dell'Aula, per rappresentarle quanto segue. È da più di venti giorni che, insieme ad altri tre colleghi, abbiamo chiesto alla Presidenza il riconoscimento... PRESIDENTE.

di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo Draghi il 30 aprile scorso, si articola, come è noto, in sei missioni: digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute.

Inoltre, in coerenza con le strategie trasversali per il riassorbimento dei divari di genere, generazionali e, in questo caso, territoriali, oltre il 40 per cento delle risorse territorializzabili sono destinate al Mezzogiorno.

ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare approvato dall'articolo 1, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso Il Fondo complementare prevede 30 progetti, di cui 20 sono già previsti e cofinanziati con il PNRR, mentre 10 progetti sono completamente nuovi e finanziati dal Fondo complementare. In ogni caso, tutti e 30 i progetti rispondono alle linee guida e agli obiettivi previsti dal PNRR. Il provvedimento in conversione si compone di sei articoli, dei quali l'articolo 1 tratta appunto del Piano nazionale per investimenti complementari, finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per - lo ripeto - 30,6 miliardi per gli anni dal 2021 al 2026. Il comma 2 prevede di ripartire il fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo profilo finanziario annuale per ciascuno delle annualità citate. In particolare, gli interventi finanziati con il Fondo complementare

ulteriormente potenziati da un emendamento e da un ordine del giorno approvati in Commissione; 9.760 milioni destinati al Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili per il rinnovo delle flotte, il rafforzamento delle linee regionali, il rinnovo del materiale rotabile, il programma Strade sicure, il monitoraggio dinamico per il controllo remoto di ponti, viadotti e tunnel, lo sviluppo e l'accessibilità marittima dei porti, l'elettrificazione delle banchine e le aree interne. Si tratta e alcuni sono stati potenziati sia da emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, sia da ordini del giorno che impegneranno il Governo a intervenire nei prossimi provvedimenti, a partire dalla legge di bilancio. inoltre, 1.455 milioni per il Ministero della cultura per un piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Sono necessari 2.387 milioni per il Ministero della salute per dei programmi di prevenzione, protezione e

risorse al Ministero della giustizia per il miglioramento della situazione carceraria, con particolare riferimento alle strutture penitenziarie sia per adulti che per minori;

risorse al Ministero dell'interno per i piani urbani integrati e 4.500 milioni per la misura del superbonus. La misura del superbonus è stata ulteriormente prorogata: per quanto riguarda gli Istituti autonomi case popolari al 30 giugno 2023,

il Governo a intervenire per potenziare ulteriormente questa misura; allo stesso modo, molti degli emendamenti e ordini del giorno presentati dai colleghi in Commissione bilancio hanno raccomandato al Governo di prorogare e ampliare l'ambito soggettivo di tale intervento. A tal proposito, è da valutare molto positivamente l'articolo 1, comma 5, che vincola eventuali risparmi di spesa monitorati sulla misura del superbonus alla proroga del termine di fruizione dell'agevolazione.

di semplificazione, accelerazione e revoca delle risorse per mancato rispetto dei cronoprogrammi e mancata alimentazione dei dati che servono alle strutture di monitoraggio. adotterà un decreto per disciplinare nel dettaglio il monitoraggio e il cronoprogramma degli investimenti. A tal proposito, è utile specificare che i

dell'articolo 1, che è quello di incrementare la capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni e accelerare la realizzabilità delle opere al fine del raggiungimento degli obiettivi strettamente connessi all'ottenimento dei contributi finanziari dell'Unione europea (prestiti e sovvenzioni). L'articolo 1, comma 8, prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia preventivamente soggetta all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Inoltre, un emendamento approvato in Commissione che alle amministrazioni sia richiesto il pieno rispetto del principio dell'assenza di danno significativo agli obiettivi ambientali. L'articolo 1, comma 9, reca le misure di copertura finanziaria.

lo sforzo congiunto di Governo e Commissione bilancio (ringrazio anche tutti i tecnici) ha permesso di approvare in Commissione delle significative norme sia ordinamentali, sia onerose a valere sulla copertura della programmazione del

l'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031, secondo la seguente ripartizione: 850 milioni per il 2022, 1.000 milioni per il 2023, 1.250 milioni per il 2024, 2.850 milioni per il 2025, 3.600 milioni per il 2026, 2.280 milioni per il 2027, 2.200 milioni per il 2028, 600 milioni per il 2029, 500 milioni per il 2030 e 370 milioni per il 2031. Tale rifinanziamento si aggiunge ai 50 miliardi complessivi già stanziati dalla legge di bilancio 2021 e destinati esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese. Ne consegue, come confermato dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 2.1, che esplicita la finalizzazione dell'incremento delle risorse all'accelerazione del loro utilizzo e alla realizzazione degli investimenti previsti nel PNRR, quanto indicato dal Governo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel quale è annunciato un anticipo della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo un principio di complementarità e di addizionalità delle risorse. In particolare, secondo quanto esposto nel PNRR, la programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 verrà anticipata per un valore di circa 15,5 miliardi, per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti. Tali risorse, si sottolinea sempre nel Piano, saranno reintegrate nella disponibilità del fondo, così da garantirne la piena addizionalità.

e destinate ai territori nel rispetto della chiave di riparto dell'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del restante 20 per cento alle aree del Centro-Nord, di cui al medesimo comma 178. Le assegnazioni saranno inoltre disposte nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e le conseguenti erogazioni saranno contenute alle relative disponibilità di cassa. Durante i lavori di Commissione sono state approvate diverse proposte emendative, con le quali sono stati aggiunti i seguenti ulteriori investimenti per complessivi 700 milioni di euro: 135 milioni di euro complessivi nel triennio 2022-2024 per la realizzazione di un'unica rete di interconnessione nazionale dell'istruzione, che assicuri il coordinamento delle piattaforme dei sistemi dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero, l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette; 70 milioni di euro complessivi nel triennio 2022-2024 per la costituzione di un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire piattaforme *oil & gas* e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, in cui eolico, *off-shore* e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno contemporaneamente in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi; 300 milioni di euro complessivi dall'anno 2021 all'anno 2024 in favore dei Comuni con popolazione da 50.000 a 250.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano, nell'ottica della transizione verde, della rigenerazione urbana e sostenibile e all'inclusione sociale. Nel triennio 2022-2024, a investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria, visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili PM10 e dei valori limite relativi al biossido di azoto, di cui alla procedura di infrazione n. 2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello stretto di Messina;

estensivi e pascolivi, come all'allevamento all'aperto *grass-fed* e quello biologico per la transizione a sistemi senza gabbie. Tali risorse sono assegnate dal CIPESS, previa intesa con le Regioni, con le modalità e nel rispetto della percentuale di riparto territoriale stabilite dalla legge di bilancio 2021. L'articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 1, 1065, della legge di bilancio 2021 riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese, di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). Appare opportuno rammentare come la legge di bilancio 2020, (articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019) in luogo di prorogare al 2020 il cosiddetto superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese - misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per la specifica categoria di investimenti ha sostituito tali strumenti con un credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2020. La legge di bilancio 2021 ha poi individuato i beneficiari del credito di imposta nelle imprese che, a decorrere dal 19 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 qualora il relativo ordine sia stato accettato e vi sia stato il pagamento di almeno il 20 per cento del prezzo entro il 31 dicembre 2022 - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La modifica di cui al presente articolo si rende necessaria poiché la misura agevolativa in questione, non essendo ritenuta idonea dalla Commissione europea a contribuire in maniera efficace e significativa all'obiettivo della transizione ecologica del Paese, non può trovare copertura finanziaria nelle risorse del Next generation EU, come era stato invece previsto in legge di bilancio 2021, e vi si deve provvedere dunque con risorse proprie dello Stato italiano. In particolare, si segnala come sia la copertura prevista dalla legge di bilancio 2021 che quella posta dalla presente norma a valere sulle risorse previste dall'articolo 5, prevedono la sola copertura in termini di saldo netto da finanziare, in quanto, come riportato dalla relazione tecnica, l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto è già considerato nelle previsioni tendenziali del conto delle pubbliche amministrazioni del Documento di economia e finanza del 2021, tenendo conto dell'impatto peggiorativo sull'indebitamento netto del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento) disposto dall'articolo 1, commi 1051-1065, della legge di bilancio per il 2021. L'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria alta velocità-alta capacità Vicenza-Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Si tratta di interventi complementari a quelli previsti nel PNRR, in quanto i due lotti del completamento della tratta Vicenza-Padova, previsti al comma 1, appaiono in sinergia con l'investimento di 3,6 miliardi di euro per la tratta Brescia-Verona e Verona-Bivio Vicenza, nell'ambito delle nell'ambito delle linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa. D'altra parte, lo stesso investimento previsto al comma 2 sulla tratta alta velocità Salerno-Reggio Calabria, accompagna l'intervento previsto nel PNRR nell'ambito dei collegamenti finanziari.

ritenuto dal Governo, sin dall'avvio del suo percorso in Senato, non meritevole di un approfondito esame

In termini di contenuti invece, il decreto-legge n. 59 è piuttosto snello, essendo composto di soli 6 articoli del valore complessivo di 30,6 miliardi di euro. Tuttavia esso si si presenta con numerose lacune che emergono anche dai *dossier* redatti dal Servizio del bilancio del Senato, organo che non è certo espressione della minoranza. È singolare che persino il *dossier* che accompagna il provvedimento rilevi come anche il Parlamento non sia stato messo nelle condizioni di poter operare concretamente. Nei commenti all'articolo 1, comma 5, si rileva infatti che le Commissioni parlamentari sono destinatarie di comunicazioni relative agli aggiornamenti delle stime inerenti il superbonus; comunicazioni che vengono definite dai tecnici che hanno redatto i documenti come mere informative, mentre invece viene suggerito nel testo stesso, di valutare: «l'opportunità di accompagnare l'aggiornamento delle stime con una relazione tecnica e prevedere in proposito l'espressione di un parere parlamentare». In pratica anche i tecnici notano che il Parlamento è stato relegato al ruolo di spettatore rispetto alle decisioni del Governo. È singolare quanto riportato rispetto ai contenuti dell'articolo 3, relativo ad ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0. L'analisi nota che sebbene l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, è già considerato nelle previsioni tendenziali del Documento di economia e finanza «occorre dare riscontro circa l'impatto di ogni singola disposizione, non potendo ritenersi sufficiente la generica rassicurazione che la misura è già stata inclusa nelle previsioni tendenziali senza che ne sia fornita separata evidenza». In pratica si è giocato con i numeri. Concetti simili sono riportati anche rispetto all'articolo 4, relativo agli interventi di finanziamento in materia di linea ferroviaria ad alta velocità, inerente in particolare la linea Verona-Padova e la linea Salerno-Reggio Calabria. Rispetto a questi interventi mancano i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere; pertanto, anche in questo caso, pur trattandosi di investimenti limitati, non risulta ancora possibile una valutazione esaustiva in tal senso. I tecnici del Senato rilevano altresì che non risulta possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto per gli anni successivi al 2024. Anche in tal caso mancano alcune valutazioni. È però all'articolo 5 che bisogna prestare attenzione perché quel che si evince leggendo i *dossier* di documentazione è che per gli oneri da finanziare per l'anno 2021 mancherebbe una copertura pari a 50 milioni di euro, in quanto gli articoli 1, 3 e 4 stimano oneri pari a 6,340 miliardi che diventano 6,290 miliardi nel citato articolo 5. Dove li prenderemo questi 50 milioni mancanti o dove li perderemo non è dato saperlo e questo qualcuno del Governo dovrà anche spiegarcelo. Capiamo che su 6 miliardi di spesa, 50 milioni sono meno dell'un per cento, ma in tempi di crisi anche l'un per cento di risorse può fare la differenza e comunque una svista da 50 milioni di euro denota l'attenzione con la quale la maggioranza cura i provvedimenti con cui dice di voler risollevare Italia. Come minoranza abbiamo presentato emendamenti migliorativi, alcuni dei quali potevano trovare una copertura semplicissima abolendo il *cashback,* miliardi di euro buttati.

ma probabilmente Governo e maggioranza ritengono che Roma sia da trattare alla stregua di un capoluogo di provincia. Infine, per onestà intellettuale è doveroso ammettere che, se c'è un provvedimento giusto assunto dal precedente Governo Conte II, questo provvedimento prende il nome di superbonus. Tuttavia, abbiamo più volte segnalato in tutte le sedi come la complessità della procedura burocratica, unita alla scadenza fin troppo breve, rendano la misura poco praticabile e poco credibile. Anche questa volta abbiamo chiesto una sua proroga fino al 2023, ma anche in questo caso constatiamo che gli emendamenti in tal senso sono stati tutti bocciati dalla maggioranza, rischiando di vanificare gli effetti di una misura tanto attesa quanto impraticabile, stanti gli stringenti vincoli legati in particolare alla durata. In conclusione, signor Presidente, viste le criticità che ho elencato, c'era un ampio margine per migliorare il provvedimento, se solo il Governo non si fosse chiuso in se stesso: ciò fa sì che quest'Aula si debba per l'ennesima volta misurare con un provvedimento molto lacunoso.

il senatore Calandrini, che mi ha preceduto, ha chiaramente esposto le ragioni che non piacciono a Fratelli d'Italia e che ci hanno visto critici, non tanto e non solo nei contenuti, ma soprattutto nel metodo, a proposito del tema PNRR e quindi naturalmente anche del cosiddetto "fondone" complementare. Riteniamo che il Parlamento avrebbe dovuto avere un ruolo maggiore di quello al quale viene invece demandato: avrebbe dovuto poter discutere e collaborare di più con il Governo, cosa che invece non accade purtroppo Non dimentichiamo, colleghi, che anche questo provvedimento vale una buona finanziaria del tempo passato, un provvedimento da oltre 30 miliardi di euro, che è arrivato nelle Aule parlamentari quasi stancamente, trascinando maggioranza e opposizione senza quasi sapere quando lo avremmo dovuto trattare: fino a questa mattina neppure eravamo certi di esaminare questo decreto. Permettetemi di dire che questo comportamento - e mi rivolgo alla rappresentante del Governo e ai rappresentanti della maggioranza della maggioranza - non è rispettoso verso la democrazia parlamentare che noi vogliamo tutelare in ogni giorno della nostra attività. Detto questo - e mi sembrava importante ribadirlo - approfitto della valenza e del significato di una discussione generale per inquadrare il tema del PNRR e del fondone complementare. Vogliamo farlo innanzitutto perché solamente se saremo in grado di garantire le condizioni migliori per l'efficienza e l'efficacia dei provvedimenti, potremo dare al nostro Paese delle prospettive di seria e stabile ripresa.

Paese caratterizzato solamente per il sospetto, per il giustizialismo, per la cultura di incriminare chiunque avesse la voglia e il coraggio di fare e soprattutto il coraggio, talvolta, di accorciare le procedure. Se vogliamo garantire al sistema Paese una efficacia davvero totale, dobbiamo semplificare ovunque.

per poter fare interventi di questo tipo, quindi la proroga doveva essere immediata, anzi era già in ritardo, avreste dovuto farla già prima. quindi disatteso una richiesta non ideologica, non di parte, ma di buonsenso, che veniva dalle imprese, dagli utilizzatori, da coloro che devono utilizzare, per il bene del Paese, il superbonus 110

che devono portare il Paese verso la sostenibilità del proprio sistema produttivo. Siamo tutti d'accordo che si tratti di un'iniziativa interessante ed importante. Anche su questo, permettetemi una chiosa. Prima di tutto, vorrei chiedere al Governo di capire meglio dal Ministero dello sviluppo economico le ragioni, veramente indecifrabili e incomprensibili per chi fa impresa, del fatto che la cosiddetta fondazione Neatech starebbe per cambiare nome in fondazione Medical. Al di là dei nomi, questo vuol dire, signori della maggioranza e signori del Governo, che nell'ambito di questo percorso si rischia di vanificare le attese di molte imprese italiane nel settore delle *startup.* Quello che voglio dire è che su questi temi abbiamo bisogno di assoluta chiarezza, di dare risposte al nostro Paese. Concludo con un altro aspetto fondamentale, quello della cessione dei crediti di imposta. Anche su questo Fratelli d'Italia ha preparato un'interrogazione. Dobbiamo sostenere la trasferibilità dei crediti d'imposta: è inaccettabile, signori, che Eurostat voglia condizionare, per la Transizione 4.0, la cessione dei crediti d'imposta, considerandoli come crediti pagabili.

nel momento in cui vengono utilizzati, cioè nei cinque anni, le entrate fiscali dello Stato, a fronte di retroazioni fiscali ben più importanti, che sviluppano l'economia. Non è quindi ammissibile che il Governo accetti passivamente questa classificazione. Dobbiamo dare impulso alla cessione dei crediti di imposta; dobbiamo dare impulso alla moneta fiscale, perché è uno strumento

Per concludere, signor Presidente, mi permetta di condividere le preoccupazioni e le sollecitazioni della neo presidente di Assonime, che ha detto chiaramente quanto ho cercato di dire io nel mio intervento: non vanifichiamo la riuscita del PNRR e del fondone, quindi implementiamo

più coraggio, perché davvero i soldi che investiamo nel nostro Paese possano garantirci quello sviluppo necessario affinché possiamo uscire finalmente da questa difficile situazione di crisi.

siccome condivido la relazione di maggioranza portata in Assemblea dalle senatrici Rivolta e Conzatti, mi soffermerò rapidamente su un aspetto che è rimasto decisamente in ombra, quando parliamo di Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un investimento mastodontico ed è risaputo che richiede al contempo rapidità, trasparenza e coinvolgimento. Si è giustamente lavorato sul lato della semplificazione, però ci si è dimenticati di lavorare per generare un rapporto più equilibrato tra organi dello Stato. La gestione del *recovery fund* è destinata, infatti, a riscrivere i rapporti tra Governo e Parlamento ed è destinata, a sua volta, a rivisitare i rapporti all'interno del Governo, prevedendo un'evidente centralizzazione attorno al Presidente del Consiglio dei ministri. È una sorta di ritorno al tempo delle piramidi, dove alla verticalizzazione del potere corrisponde una base decisamente più larga e quindi meno coinvolta. La marginalizzazione del Parlamento, signor Presidente e Governo, ha una causa legata alla riduzione del numero dei parlamentari. Sappiamo già oggi che il Senato avrà difficoltà a lavorare al meglio in questa condizione, salvo che divenga una Camera diversa da quella che è, ossia una Camera di solo controllo o una Camera delle autonomie. Sappiamo anche che questa condizione non è raggiungibile nel corso di questa legislatura. La domanda che dobbiamo porci, accanto all'aspetto economico e di gestione finanziaria del Piano, è come si innesti la cabina di regia del Governo sul *recovery plan* contestualmente, sull'attività parlamentare e, quindi, come si possano esaltare le funzioni di proposta e di controllo delle Camere riguardo un piano di investimenti che non ha uguali nella storia recente della nostra Repubblica, salvo riandare con la memoria al piano Marshall di diversi anni fa. La mia opinione è che la linea di condotta vada tracciata ora proprio perché vige un rapporto di unità nazionale nel Governo dell'Italia. Il Piano, infatti, insisterà per un po' meno della metà su questa legislatura e per più di metà sulla prossima legislatura, presumibilmente, avrà caratteristiche diverse da questa. Passeremo dall'unità nazionale, molto probabilmente, a due o più schieramenti che si confronteranno con gli elettori che sceglieranno chi dovrà sedere sui banchi del Governo e chi dovrà sedere tra i banchi dell'opposizione. Ragione in più per fissare oggi le regole di ingaggio, oggi che inizia un percorso di questa natura. è di dedicare una seduta parlamentare alla discussione del futuro dell'Italia visto da questa parte, visto cioè da questa angolazione, da questo osservatorio. Già qualcosa, attorno a noi e fuori da noi, si muove e noi lo valutiamo in maniera assolutamente positiva. Dal G7 si intuisce un'attenzione maggiore al quadro geopolitico. L'Europa prova a riconquistare un ruolo di centralità in un rapporto euro-atlantico, che era stato decisamente accantonato.

Si sostiene la tesi della funzione storica delle democrazie e, quindi, anche l'Italia si appresta a costruire e a darsi una visione strategica, che è destinata, da una parte, a cambiare il profilo dell'Italia medesima e, dall'altra, a giocare un ruolo che negli ultimi anni l'Italia non era assolutamente solita ricoprire. Ad un anno e mezzo dalla fine della legislatura e con in mezzo l'elezione del Presidente della Repubblica, trovo poco realistico parlare di riforme costituzionali. Non di meno, se non si parla di riforme costituzionali, è obbligatorio invece immaginare un sistema equilibrato, che definisca meglio i rapporti fra legislativo ed esecutivo. una seduta parlamentare, quindi, che affidi ad una risoluzione un indirizzo, rivolto intanto al Senato, affinché le due Commissioni affari istituzionali di Camera e Senato, oppure una Commissione speciale ristretta, con tempi ben definiti,

il procedimento legislativo, perché il Parlamento, con le sue Commissioni, non venga messo da parte a partire dal governo del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ad una Costituzione materiale, signor Presidente, deve corrispondere perlomeno un equilibrio materiale tra poteri dello Stato, come ci ricordava Costantino Mortati.

oggi non sono più in grado di farlo, noi non possiamo attendere che sia la Corte costituzionale a definire il percorso: sia il Parlamento allora ad avviare questa soluzione. Che non si dica, come troppi anni fa, che il Parlamento si presenta al Governo e non viceversa.

Mi prende qui ringraziare per il lavoro svolto in Commissione dalle relatrici Conzatti e Rivolta perché si è lavorato molto bene.

non c'è grande soddisfazione per il percorso - non per il contenuto - né per la modalità; abbiamo assolutamente bisogno che venga rivisto il *modus operandi*, perché riuscirà difficile nel prosieguo che si possa arrivare a conclusioni condivise. Il provvedimento contiene tanti punti: alcuni riguardano interventi di finanziamento sulle linee ferroviarie ad alta velocità e alta capacità, che riguardano per lo più il Nord-Est e la tratta Salerno-Reggio Calabria; c'è

italiani in povertà assoluta: attenzione, perché la bomba sociale prima o poi scoppia. Dobbiamo fare le riforme, farle in fretta e bene. Il Governo, con l'autorevole Presidenza del presidente Draghi,

Signor Presidente, signori senatori, il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021 reca misure urgenti relative al fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti; si pone l'obiettivo di integrare di integrare la dotazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza con ulteriori risorse nazionali per oltre 30 milioni di euro. Il testo della norma prevede diversi interventi, tra cui stanziamenti per lo sviluppo della mobilità sostenibile e dei trasporti ferroviari ad alta velocità. A questi si affiancano nuove dotazioni per il MIC destinate allo sviluppo turistico e alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico. A tali misure si aggiunge un incremento della dotazione del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, pari a 15,5 miliardi di euro. Ciò per colmare le differenze di sviluppo tra i territori che rallentano la crescita e ostacolano il progresso, soprattutto al Sud Italia. La ripresa dell'Italia non può prescindere dalla piena valorizzazione culturale ed ambientale delle bellezze che caratterizzano tutti i nostri territori. Assicurare una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale vuol dire garantire facilità nell'accedere e nel raggiungere i siti archeologici, i luoghi di interesse artistico e paesaggistico. A tal proposito ricordo che il decreto-legge cosiddetto fondone interviene autorizzando una spesa per oltre 9 miliardi di euro affinché sia realizzata l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, con il fine di superare i limiti infrastrutturali esistenti. La provincia di Salerno, ad esempio, che mi pregio di rappresentare, è ricca di cultura e trabocca di tesori archeologici e di beni paesaggistici e artistici; luoghi meravigliosi, che scontano però una grave insufficienza delle reti di collegamento, cosa che finisce per soffocarne le potenzialità turistiche e le occasioni di sviluppo. L'alta velocità, pur rappresentando un'opera indispensabile, non è purtroppo risolutiva dei problemi di collegamento che affliggono questi territori ricchi di storia, di bellezza e di prodotti enogastronomici di eccellenza. Il tema mi è molto caro e per questo ho presentato un emendamento e un ordine del giorno, affinché il Governo valuti la possibilità di affiancare alla nuova alta velocità una metropolitana di superficie che possa collegare i siti archeologici dei Comuni dell'entroterra. Si pensi, ad esempio, al Vallo di Diano o ai luoghi meravigliosi della certosa di Padula e delle grotte di Pertosa, che scontano la totale assenza di collegamenti ferroviari e che sono serviti solo da trasporto su gomma. I Comuni di Pertosa e di Padula saranno attraversati dalla futura linea alta velocità, ma questa non contempla alcuna fermata intermedia presso tali siti. Per tale motivo sono convinta che sarebbe auspicabile si realizzasse con l'occasione anche una nuova linea che affianchi i binari dell'alta velocità. Collegando le aree interne si risolverebbero i gravi *deficit* di trasporto ferroviario che gravano su questi luoghi. Inoltre, ho proposto di realizzare una stazione ferroviaria presso l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, dove sono previsti lavori di ulteriore allungamento della pista, proprio al fine di incentivare i collegamenti turistici non solo in Campania, ma anche per le Regioni confinanti come la Calabria e la Basilicata. L'aeroporto, pur trovandosi in prossimità della tratta ferroviaria che collega, ad esempio, l'antica città di Paestum e il sito archeologico di Elea-Velia, non è dotato di una stazione che permetta l'accesso dei viaggiatori alla linea ferroviaria già esistente esistente e attiva. Credo che sia indispensabile rimediare; i vantaggi sarebbero a questo punto incalcolabili. La stazione ferroviaria in prossimità dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, infatti, permetterebbe ai turisti di accedere comodamente alla costa cilentana e alla costiera amalfitana, nonché alle aree interne e al porto di Salerno, con costi e impatto ridotti al minimo e con benefici che produrrebbero effetti positivi ben oltre la provincia, andando a favorire i collegamenti in buona parte del Sud Italia. Questo provvedimento ci offre l'occasione per colmare un po' delle differenze negative che il nostro Paese sconta in termini di infrastrutture. Madre natura con questi territori è stata molto generosa e materna; il resto lo ha fatto la storia. A noi resta la responsabilità morale e politica di valorizzare

rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, oggi ci apprestiamo ad approvare il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Questo provvedimento è finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR stesso; le risorse aggiuntive sono pari a 30,6 miliardi per gli anni dal 2021 al 2026, che si vanno a sommare ai 204,5 miliardi previsti dal PNRR, ai quali l'Italia ha potuto accedere grazie ai programmi Recovery and resilience facility e React-EU. La somma totale dei due interventi corrisponde a 235 miliardi circa. Queste risorse sono necessarie per il rilancio dell'economia nazionale, che risulta tra le più colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. È evidente che bisogna essere consci di quale tipo di modello di sviluppo vogliamo per il nostro Paese. È opportuno avere ben chiari quali sono i nostri obiettivi per uno sviluppo sociale ed economico, in quanto la visione avrà ripercussioni per gli anni a venire. Saremo i decisori del futuro delle prossime generazioni e non possiamo permetterci di sbagliare, non più. Non possiamo permetterci di avere una visione miope; non possiamo permetterci di rimanere indietro rispetto agli altri Paesi europei. Sicuramente una delle cose che dobbiamo fare è un'analisi di cosa ci ha reso vulnerabili in questo periodo di pandemia, che ha sottolineato tutte le criticità delle scelte politiche passate. L'urgenza di tutelare la nostra salute da nuovi e sconosciuti mali ha ribadito l'importanza della ricerca scientifica e dell'utilizzo della tecnologia - diventata in quest'ultimo anno fondamentale per lo svolgimento delle attività lavorative, per lo studio e per connettere le persone - e la necessità e l'urgenza di restituire alla natura la sua dignità, ripensando anche al consumo del suolo e all'inquinamento, e di ridare pari dignità a tutti i territori, creare nuove infrastrutture per connettere i centri con le zone marginali. Insomma, bisogna ricostruire il benessere sociale ed economico dei cittadini. Questo è il ruolo della politica, che deve tornare a educare e proporsi come strumento formativo di stili di vita e perché ciò avvenga deve avvicinarsi alla gente, alla quotidianità delle cose e non deve perdere di vista la realtà nella sua concretezza. Per questo i finanziamenti del Piano di ripresa e resilienza devono essere attuati e realizzati anche attraverso il protagonismo delle Regioni, delle Province e dei Comuni. L'Italia, proprio per la sua bellezza, è uno dei Paesi più invidiati al mondo, perché racchiude in sé tutto ciò che uno Stato può desiderare: con le sue isole è circondata dal mare, ha un'estensione montana (le Alpi e gli Appennini) e la pianura Padana. territori diversi tra loro, che devono però trovare le adeguate risposte proprio per le specificità che li distinguono. Tra i temi affrontati sia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia nel Fondo complementare vi sono i seguenti: mettere in connessione i territori, investendo in nuove infrastrutture, nella creazione e nel rafforzamento rafforzamento dei servizi in ambito sanitario e assistenziale; puntare su un'economia *green*, partendo proprio dal risparmio energetico e dalla mobilità sostenibile con l'implementazione e il rinnovamento delle flotte degli autobus, con mezzi più ecologici; potenziare le ferrovie regionali, collegando con porti e aeroporti; intervenire sull'ammodernamento delle reti di distribuzione idrica, sulla messa in sicurezza e sull'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel; migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade, senza consumo di suolo, aumentando la resilienza a fenomeni sismici e dissesto idrogeologico. Quando ci riferiamo alla mobilità sostenibile, è evidente che parliamo anche di nuove ciclovie. Sarebbe importante valutare investimenti su trasporto a fune, collegando i paesi a valle con la montagna. Questi investimenti hanno valenza di trasporto alternativo, decongestionando il traffico sulla strada, migliorando sia la qualità della vita degli abitanti sia quella dell'ambiente.

Per fare ciò è evidente che bisogna tenere in piedi e aiutare le piccole e medie imprese, mettendo in campo non solo investimenti, ma anche riforme, partendo dalla semplificazione e dalla riforma della giustizia e fiscale. Gli investimenti previsti dai due provvedimenti aiuteranno anche a creare occupazione, ma credo sia importante in questo momento investire ulteriormente sulla riduzione del cuneo fiscale e sul lavoro per incoraggiare l'assunzione e ridare potere d'acquisto ai lavoratori.

ai polimeri, ai metalli industriali, a rame, nichel, acciaio e alluminio), nonché dei semiconduttori. Questa carenza porta all'incremento dei prezzi, determinando l'annullamento e la rinegoziazione delle commesse, generando problemi alle aziende sui lavori già messi a dura prova dalla pandemia.

innovativo, ma anche costruttivo e sicuramente utile una parte delle risorse destinate allo sviluppo e alla coesione. Ciò è stato fatto con il permesso delle Regioni ed è stabilito che

E se nella scuola non inseriamo strumenti innovativi affinché migliorino il servizio scolastico, nonché la connessione tra le scuole, l'Ufficio regionale scolastico e il Ministero, non potremo mai ottenere un servizio all'altezza.

quello che ci apprestiamo ad approvare oggi è un atto importante, con cui entriamo finalmente nel vivo rispetto a due principi e due spinte che ci hanno animato negli ultimi mesi: da un lato, il PNRR e, dall'altro, si è aggiunto

sicuramente una valenza relativa all'ambiente. È chiaro che l'inclusione sociale passa per il ripensamento e la progettazione delle nostre città, in particolare delle periferie, e questo non può che avere anche una valenza di carattere ambientale, che si incrocia con un percorso peraltro avviato in questi tre anni relativamente

perché dà concretezza a una visione di fondo. Lo stesso potrebbe dirsi anche per l'impostazione che anima la Lega. In questo caso, se da un lato lo sviluppo edilizio degli anni Sessanta e Settanta ha lasciato tracce indelebili pesantissime e ferite ancora aperte nelle nostre città, non è bloccando e cristallizzando tutto che si può porre rimedio a quell'errore; non è come in matematica, in cui meno per meno fa più, perché due quindi, non è un accanimento nell'individuare una soluzione, ma vuol essere la risposta che permetta agli imprenditori illuminati, alle amministrazioni comunali e alle Regioni di immaginare e di avere gli strumenti per realizzare qualcosa di diverso.

di Francesco Rosi, del 1963. Ebbene, chi investe oggi in edilizia e ci crede veramente non è come Edoardo Nottola, il protagonista senza scrupoli di quel film, ma qualcuno che vuole investire e crede nella possibilità di tutelare l'ambiente e di avere uno sviluppo anche facendo impresa. Per questo pensiamo a determinate azioni e a determinati strumenti e non a caso vorremmo che il superbonus al 110 potesse essere esteso anche alle strutture ricettive, agli alberghi, ma anche - perché no - agli agriturismi, che peraltro, nel caso delle strutture ricettive, sono fra gli edifici a maggior dispersione termica e con necessità di efficientamento energetico, per risolvere anche il problema della dispersione di calore. Questo è un tema. Avviandomi alla conclusione, è quello relativo agli eventi sismici. Aver individuato 1,780 miliardi per gli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel 2009 e nel Centro Italia nel 2016 è sicuramente meritorio. riteniamo (e per questo abbiamo presentato un ordine del giorno) che sia importante inserire anche gli eventi sismici dell'Emilia del 2012, ma la cosa fondamentale, su cui chiediamo uno sforzo, è cambiare impostazione.

oggi abbiamo dovuto individuare 100 milioni, potrebbe succedere ancora. Pertanto, l'appello che rivolgo al Governo in conclusione è anche di dare per una volta attuazione a qualche ordine del giorno, in particolare a quello a mia prima firma della Lega, che chiede l'istituzione dell'osservatorio permanente sulla ricostruzione (OPR), andare a vedere, di tutte le risorse impiegate e investite dal terremoto dell'Irpinia del 1980 ad oggi, cos'è stato effettivamente fatto e cosa ancora manca, perché è inutile fermarsi alle buone intenzioni e metterci anche le risorse, se poi non siamo in grado di attuare quello che ci proponiamo.

individuando i programmi e gli interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse tra gli stessi, per singola annualità. Per ogni misura è individuata l'amministrazione competente. Nell'analisi del testo ho avuto modo di notare quanto già premesso dal collega Briziarelli, ossia all'articolo 1 la destinazione di 1,78 miliardi ai territori colpiti dal sisma. Nell'articolo vengono considerati i sismi del 2009 e del 2016. Nella Commissione bicamerale sulle questioni regionali è stato votato un parere inserendo il sisma del 2012; ma alla richiesta dell'inserimento del sisma 2018, il cosiddetto sisma di Santo Stefano, che ha colpito nove Comuni della Provincia di Catania,

del 2018, oltre a quello del 2012. La ringrazio perché quest'ordine del giorno, che nel gergo parlamentare sembra un qualcosa di poco significativo, in realtà assume un significato importante proprio in questo momento storico, perché noi ci apprestiamo al semestre bianco. Il semestre bianco sarà il semestre dell'oblio?

ho assistito personalmente, anche al tavolo di lavoro allora presieduto da Curcio, a un lavoro che doveva essere congiunto, includendo l'intervento per i sismi in tutto il territorio italiano, ma puntualmente così non è stato. Puntualmente la Sicilia viene sempre dimenticata le giustificazioni sono sempre le solite, come se i governatori siciliani, o comunque chi è preposto, fossero inadeguati o non avessero una gestione del denaro soddisfacente

si è data rilevanza solo al terremoto dell'Aquila? Sono dodici anni che assisto a fiumi di denaro. Nel mio caso la mia casa è stata plurifinanziata; pensi che è stato pagato l'architetto che ha redatto il progetto con circa 300.000 euro,

Poi è arrivato un sindaco che nel 2017 ha operato la demolizione, ma di ricostruire non se ne parla. Mi viene negato accesso agli atti per ben due volte; non mi danno riscontro neanche per un alloggio equivalente. Io che cittadina di serie sono? Di serie A o B? Sicuramente di serie H, a riprova del fatto che tale narrazione distorta di un Sud incapace di gestire deve finire. Adesso il Governo si è assunto l'impegno di provvedere alla ripartizione dei fondi anche per il sisma nella provincia di Catania, che è stato, sì, finanziato fino al 2023, ma la destinazione del fondo di riferimento è fino al 2026 e i fondi già stanziati non saranno sicuramente sufficienti. Altro argomento che mi preme evidenziare il famoso tema del Ponte sullo Stretto. Come sapete, è stato creato un intergruppo su di esso. È stata data visibilità ad Italia viva e Forza Italia. Devo dire, con sommo rammarico, che non si è tenuto conto del parere condizionato del Vice Presidente della Regione siciliana durante la Conferenza Stato-Regioni del 3 giugno, in cui auspica assolutamente l'intervento e l'imprescindibilità della relazione del Ponte sullo Stretto, da inserire quindi nel PNRR. Non solo non si è data visibilità, ma addirittura

l'implementazione della flotta navale, quindi l'attraversamento dello Stretto, e la rigenerazione urbana sostenibile - guarda caso di Reggio Calabria e Messina. Concludo dicendo che siamo tutti servi inutili e che nella prossima legislatura non è certo che le persone che risiedono in questi scranni saranno nuovamente qui presenti. Noi siamo chiamati a lavorare per gli italiani.

certamente provati, ma diversi. Sono già cambiati e cambieranno ancora tanti costumi e modi di operare e anche di lavorare. Penso alla diffusione dell'uso delle piattaforme per le videoconferenze, alle quali ormai ci siamo abituati. Occorre dare corso a riforme anche importanti ed è nostro dovere operare per correggere le storture che hanno fermato la crescita di questo Paese. È venuto il momento di ricostruire, cambiare, rimboccarsi le maniche, agevolare e non ostacolare chi lavora, le nostre piccole e medie imprese, *in primis*, ma anche quelle grandi, per una spesa e per investimenti realmente costruttivi. Il Fondo complementare al PNRR nasce proprio per finanziare tutti quei progetti che, per loro stessa natura, non potevano rientrare nel *recovery plan* plan* e prevede investimenti che serviranno a finanziare progetti a partire da oggi e per i prossimi cinque anni. Riporto in sintesi alcune misure, di cui si è già detto, che verranno intraprese con i finanziamenti del Fondo. I primi investimenti riguardano la digitalizzazione; sono previsti per i servizi digitali e la cittadinanza digitale, le competenze, le tecnologie satellitari, gli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; vi sono ulteriori interventi destinati ai terremoti del 2009 e del 2016. Per quanto riguarda i trasporti, si interverrà nel rinnovo di flotte, di bus, treni, navi verdi, nel rafforzamento delle linee regionali, nel rinnovo del materiale rotabile, in strade sicure nell'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e gallerie. Faccio un inciso: da qualche decennio, abbiamo trascurato una tipologia di lavori che riguarda tutto il nostro patrimonio di opere storiche e anche le infrastrutture più recenti; si tratta della categoria di lavori compresi in quella che viene definita, con un sostantivo accompagnato da un aggettivo, come manutenzione ordinaria. Mi soffermo su questo concetto, perché lo ritengo assai utile. Tante volte basta un tempestivo intervento, anche esiguo in termini di costi, nella fase iniziale di un qualunque fenomeno di degrado di una qualunque opera e infrastruttura, perché questa non vada celermente in rovina, e di infrastrutture da risanare ne abbiamo tantissime, su alcune delle quali occorre anche intervenire con urgenza. previsti investimenti per il nostro incommensurabile patrimonio architettonico, storico e culturale (edifici e anche aree naturali). Ribadisco Ribadisco che nella nostra penisola e nelle nostre isole esiste e insiste uno dei più grandi patrimoni storico-culturali d'Europa e del mondo intero, che ha radici profonde e millenarie, vestigia uniche e non replicabili. Ci sono poi altri investimenti nei contratti di filiera e distrettuali per settori come l'agroalimentare, la pesca, l'acquacoltura, la selvicoltura, la floricoltura e il vivaismo. Anche qui entriamo in un contesto, quello della produzione agroalimentare, che è peculiarità unica per varietà, qualità e cultura. È previsto anche un rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione e un fondo complementare per il superbonus. È chiaro che questo *new deal*,questo nuovo corso, ha una portata storica e rappresenterà un'occasione unica in questo inizio del XXI secolo. È altrettanto evidente che serviranno strutture e apparati dello Stato, degli enti locali e di ogni organo e ufficio chiamati ad autorizzare e gestire i progetti e gli investimenti, capaci di affrontare con spirito fortemente costruttivo il processo. È un cambio di passo che dovremo affrontare con semplice pragmatismo per rilanciare uno sviluppo sostenibile mirato al rispetto dell'ambiente e, pertanto, di noi stessi e delle future generazioni. In una parola, serve responsabilità. Occorrerà lavorare, crederci e semplificare. Non abbiamo altro modo, donne e uomini di questo Paese, che quello di rimboccarsi le maniche, come hanno fatto i nostri avi in epoche anche assai più difficili, quando Luigi Einaudi affermava: «Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante

Signor Presidente, oggi quest'Assemblea ha la possibilità di intervenire nel provvedimento in discussione a tutela del benessere animale, questione assolutamente urgente e congrua con il Piano di transizione ecologica, ma purtroppo assente nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La sensibilità dei cittadini alle condizioni in cui sono allevati gli animali negli allevamenti è sempre crescente. Negli anni lo hanno dimostrato molteplici indagini, tra cui quella dell'eurobarometro nel 2016. Più recentemente, nel 2019, l'iniziativa dei cittadini europei "End the cage age", lanciata da Compassion in world farming insieme ad altre 170 organizzazione europee, tra cui 21 italiane, ha ricevuto il mio sostegno e quello di altri senatori e deputati dell'intergruppo per i diritti degli animali. Nell'Unione europea sono oltre 300 milioni gli animali (galline, scrofe, quaglie e conigli) che soffrono a causa della reclusione in gabbie anguste, che limitano severamente la loro possibilità di movimento. In Italia sono 45 milioni gli animali allevati in queste condizioni. L'iniziativa ha riscosso un enorme successo, raccogliendo 1,4 milioni di firme di cittadini europei, di cui oltre 90.000 italiani. La petizione è stata sostenuta, inoltre, da 140 scienziati, tra cui anche l'etologa e ambientalista di fama mondiale Jane Goodall; anche importanti aziende hanno pubblicamente dato il loro sostegno. A seguito di questa grande mobilitazione, proprio la scorsa settimana, il Parlamento europeo ha votato con una schiacciante maggioranza una risoluzione che esorta la Commissione europea a vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti entro il 2027, impegnandosi a sostenere gli allevatori e produttori con sussidi che favoriscano e sostengano la transizione a sistemi senza gabbie. Il commissario per la salute Stella Kyriakides ha partecipato al dibattito e ha commentato che l'impegno della Commissione per migliorare il benessere degli animali rimane un imperativo morale, sanitario ed economico. Aggiungo che non si tratta solo di una sensibilità verso gli animali, ma anche a tutela della salute pubblica, se è vero che tali metodi sono causa dell'antibiotico-resistenza negli uomini, dell'eccessiva produzione di anidride carbonica e di metano e anche, com'è stato provato, della diffusione di epidemie. La transizione verso sistemi più rispettosi del benessere degli animali, che è stata chiesta con forza e democraticamente dai cittadini italiani ed europei, è oggi quindi un'istanza di grande rilievo. Il Parlamento europeo ha ascoltato la richiesta e anche nel nostro Paese, a livello locale, le Regioni Abruzzo ed Emilia-Romagna hanno votato importanti risoluzioni in tal senso. Si registra quindi la volontà di non rimanere indietro. Per questo motivo è fondamentale oggi approvare il sostegno finanziario agli allevatori per la transizione a sistemi senza gabbie, con l'emendamento a prima firma del senatore Pesco, che al punto 3 chiede di aggiungere l'articolo 1-*bis* incentivi ad allevatori per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto. La transizione a sistemi senza gabbia è lo *standard* di più alto livello per il benessere animale, ormai inevitabile. La priorità ora è fare in modo che il nostro Paese non resti indietro e provveda con i necessari strumenti a far sì che la zootecnia italiana non subisca la concorrenza di altri Paesi europei. In tal senso, vorrei ringraziare, oltre al senatore Daniele Pesco, primo firmatario, anche il nostro capogruppo in Commissione bilancio Gianmauro Dell'Olio e il nostro ministro Stefano Patuanelli, che sta sostenendo questo importante passaggio di civiltà, etico, economico e sanitario.

ben altro dibattito, quantomeno per rispetto nei confronti dei soldi pubblici che andiamo a utilizzare. Questa è l'ennesima manovra a debito: ricordo a tutti che stiamo parlando di PNRR e di *recovery plan* come fossero la panacea e la soluzione di tutti i mali, quando questo in un anno e mezzo ha già deliberato l'utilizzo di risorse a debito per lo stesso importo, oltre 200 miliardi. A dire la verità, là fuori se ne sono accorti in pochi, anche perché il metodo utilizzato, quello dei contributi a pioggia, spesso ha segnato

a debito, dopo che per anni l'Europa invece ci aveva costretti all'*austerity.* Gli esponenti dei partiti che hanno governato fino ad oggi ci hanno sempre spiegato che ce lo chiedeva l'Europa, che ci imponeva cioè di frenare sugli investimenti, sul sociale

In questi anni lo Stato è arretrato, in nome di quell'*austerity* di cui vi siete riempiti la bocca, che ha portato a una bassa produttività delle nostre imprese e all'incapacità - purtroppo, dato proprio il sistema produttivo di questa Nazione - di cogliere le opportunità, per una mancanza infrastrutturale. È una realtà legata alle nostre piccole medie imprese, che da anni qualcuno

alla mercé di questi grandi gruppi. In realtà, le nostre piccole e medie imprese costituiscono da sempre la forza di questa Nazione, la vera biodiversità economica, altro termine di cui vi riempite la bocca, nella maggior parte dei casi senza sapere nemmeno cosa significhi

si leggano solo i titoli o le figure (se dovessero essercene). Gli investimenti in Italia sono aumentati, sempre negli stessi anni di riferimento, del 66 per cento, mentre in Europa del 118. Ecco, basterebbe questo dato per farci capire che forse quelle politiche imposte erano erano fallimentari. La quota pubblica di investimenti però è scesa dal 14,6 al 12,7 per cento, a dimostrazione di quello che dicevo, cioè che non solo si è frenato, ma si è tornati addirittura indietro.

da anni. Assieme ad esse, poi, l'Europa ci scrive anche raccomandazioni precise e puntuali, come quella di usare entrate straordinarie per la riduzione del rapporto tra debito e PIL.

che il *leader* del Partito Democratico, come prima uscita, dopo lo *ius soli*, ha pensato bene di calarla, altrimenti non riesce più a tenervi tutti uniti, se non nella richiesta di maggiori tasse (guarda caso poi gli italiani vi penalizzano, ogniqualvolta si va a votare). Ma non c'è solo questa. C'è anche la riduzione delle agevolazioni fiscali;

come la riforma dei valori catastali, un'altra patrimoniale nascosta, ancora più subdola, ma sempre presente nei vostri programmi. Poi non riuscite ad attuarla, perché perché gli italiani vi saltano sulla schiena, ma intanto la mettete sempre e ve la fate dare sempre come raccomandazione. Perché? Ce lo chiede l'Europa. Evviva l'Europa! La vostra Europa ve lo chiede; la nostra Europa, quella dei popoli, delle Nazioni e delle genti, non ha mai chiesto di stritolare l'economia delle singole Nazioni. Ha chiesto sempre di essere un'Europa dei popoli, non delle grandi multinazionali e dei burocrati, come piace a voi.

Evitiamo però di far credere cose a tutti fuori di qui, non solo a quelli che almeno una volta nella vita hanno fatto l'orto di casa, ma anche a quei tanti produttori agricoli che rendono oggi la nostra Nazione un fiore all'occhiello nel mondo delle produzioni agroalimentari. Non facciamo credere credere che la tutela dell'ambiente sia in contrapposizione con l'agricoltura, perché non è così. Dovete finire di raccontare che sono gli agricoltori a inquinare i campi. Dovete smettere di far credere alla gente che si possa sostituire la carne con quella sintetica o con le larve o con prodotti costruiti in laboratorio. *(Applausi)*. Quei prodotti non hanno nulla a che fare con la vostra e la nostra biodiversità. Noi non possiamo pretendere biodiversità quando apriamo, di fatto, alla possibilità di produrre la carne in laboratorio e abbiamo anche la supponenza di voler farle credere tale e di chiamarla carne. Non è carne! Chiamatela come volete. Mangiatevi anche le suole delle scarpe: per me non è un problema. Friggetele e mangiatevele, ma non chiamatela carne.

Certo, non ci trovate al vostro fianco quando decidete di sostituire il nostro modello di sviluppo e civiltà con un modello di sviluppo e civiltà che non ha nulla a che fare con la nostra cultura e la nostra identità, ma che è molto utile a chi vuole trasformarci in meri consumatori e in persone vuote di qualsiasi tipo di identità, perché più facilmente indirizzabili e, quindi, più facilmente schiavizzabili. *(Applausi)*.

vengono stanziate risorse importanti, che pongono le basi per una riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale che avrà, come capisaldi, la sicurezza degli edifici ospedalieri; le reti transnazionali di eccellenza, per mettere in comune competenze sia pubbliche che private e per offrire un servizio di assistenza di alta qualità; l'approccio *one health*, e cioè un nuovo assetto di prevenzione collettiva di sanità pubblica, che, con attenzione ai cambiamenti climatici e ambientali, vuole consentire una migliore promozione della salute e del benessere; gli *hub* antipandemia, con più ricerca e specializzazione dello studio per il contrasto alle emergenze sanitarie. Il cosiddetto fondone in esame destina, infatti al Ministero della salute 2 miliardi e 387,41 milioni di euro, che si aggiungono agli 8,6 del PNRR. In questa discussione merita di essere sottolineata la necessità di tornare a sostenere la sanità territoriale. Per il Partito Democratico prossimità è la parola chiave per affrontare le nuove sfide che abbiamo di fronte. Vale anche in relazione a una sanità che sia capace di essere sempre più vicina ai cittadini. Negli ultimi vent'anni, stando ai dati di Eurostat e di OCSE, sono stati ridotti di circa il 30 per cento i posti letti complessivamente disponibili negli ospedali, perché, nel corso degli anni, abbiamo dato vita a una sorta di riorganizzazione incentrata su quella che è stata chiamata la de-ospedalizzazione. Ciò che la pandemia ha messo in luce è che, a fronte di una robusta riorganizzazione ospedaliera, è mancata un'attenta riorganizzazione dell'offerta sanitaria in una visione integrata, complementare e unitaria dell'assistenza: dal medico di famiglia all'ospedale di alta tecnologia. Il punto deve essere il rafforzamento della rete territoriale delle aziende sanitarie. Le direzioni di marcia sono due: le case di comunità e l'assistenza domiciliare. Le case di comunità, però, non possono essere solo una ridenominazione delle case della salute, che a loro volta altro non sono se non la riedizione dei poliambulatori dell'INAM di parecchi decenni orsono. Si è voluto usare perché è un'idea di servizio pubblico, pur con una nuova forma di gestione sociale. Le case di comunità possono e devono essere - anche come chiedono la Caritas e altre agenzie del terzo settore - strumenti per una rifondazione del sistema di *welfare*. L'assistenza domiciliare si rivolgerà, invece, in particolare ai pazienti di età superiore ai sessantacinque anni, con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti, con l'obiettivo di aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare, fino a prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10 per cento della popolazione di età superiore ai sessantacinque anni. Questi ambiziosi progetti, Presidente, devono essere accompagnati da un riassetto del sistema ospedaliero, pensato in sinergia con quanto si deve per il territorio, e soprattutto in grado di ridisegnare complessivamente la rete nosocomiale italiana nelle sue caratteristiche e finalità e, ovviamente, proprio in virtù di quanto la pandemia ci ha insegnato, da una riorganizzazione di competenze, ruoli e funzioni tra lo Stato e le Regioni; e ciò al fine di rendere il nostro Servizio sanitario nazionale non già più efficiente da un punto di vista economico, ma più capace di rispondere in maniera adeguata alle nuove sfide sanitarie ed emergenziali che - questo lo abbiamo capito - il futuro potrà ancora riservarci.

utilizzare le risorse per colmare la disuguaglianza, anche territoriale: queste sono le condizioni di Bruxelles che hanno permesso all'Italia di accedere alla parte più cospicua del *recovery fund* rispetto a tutti i Paesi europei. Il documento della Commissione europea del 28 maggio 2020, a pagina 8, spiega quali sono i criteri per cui l'Italia ha avuto questo cospicuo fondo:

Secondo questi criteri, al Mezzogiorno, purtroppo, spetterebbe il 65 Perché questa percentuale? Basta ricalcolare la ridistribuzione adoperando gli stessi criteri di Bruxelles e, quindi, le stesse tre variabili. quindi ottenuto circa 210 miliardi solo e unicamente perché abbiamo necessità di colmare la disuguaglianza, il *gap* tra Nord e Sud, altrimenti non li avrebbe ricevuti.

cento. Chi non vuole rispettare neanche questa percentuale non vuole rispettare i criteri di Bruxelles, ma non solo. non solo. Dobbiamo ricordarci che questa è stata la precisa volontà anche del Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano. Infatti, la Camera dei deputati e il Senato si sono già espressi sul tema, chiedendo proprio l'adozione dei tre criteri di Bruxelles nella relazione sulla proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

il richiamo presente nelle linee guida del PNRR alla clausola del 34 per cento, ossia alla distribuzione dei fondi in ragione della popolazione residente, non appare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 nell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *recovery fund*, dice che appare necessario «applicare, con eventuali aggiustamenti, il criterio di riparto tra i Paesi previsto per le sovvenzioni dal Dispositivo di ripresa e resilienza (popolazione, PIL *pro capite* e tasso di disoccupazione)». Bisogna quindi usare questo criterio anche per la ripartizione tra le Regioni e le macro aree, in modo da sostenere le aree economicamente svantaggiate. Ebbene, nonostante Bruxelles ci abbia permesso di accedere a questi fondi per tale ragione e nonostante la Camera e il Senato si siano chiarissimamente espressi, neanche

Qual è il rischio? È il nodo dei progetti non territorializzati, ed è un rischio di dirottamento al Nord di ulteriori 8,7 miliardi destinati al Sud. Ormai abbiamo superato da tempo la narrativa che il Sud

investimenti statali sono sempre e comunque andati al Nord. Non possiamo permettere che questo accada

che chiede di verificare che le risorse del *recovery fund* vengano utilizzate per il riequilibrio territoriale, affinché non ci sia il rischio che i progetti non territorializzati facciano spostare gli stanziamenti ancora al Nord, per quasi 10 miliardi. Serve chiarezza nella destinazione dei fondi e quindi è necessario che, su indicazione del Parlamento, ci sia un monitoraggio della ricaduta territoriale esteso all'intero quadro del PNRR, anche al fine della verifica della legge sulla quota di investimenti ordinari da collocare nel Mezzogiorno, in proporzione

anzitutto ringraziare i colleghi della Commissione bilancio, e in modo particolare il Capogruppo, per il lavoro che è stato svolto

Quindi, la lettura dei singoli progetti, degli interventi e dei finanziamenti - secondo me - deve essere fatta inevitabilmente a specchio, perché altrimenti si rischia di perdersi in rivoli che non consentono una visione di carattere generale. Detto questo, vorrei anche ricordare che con questo provvedimento il Governo e il Presidente del Consiglio hanno adempiuto a un impegno che era stato preso con riferimento agli ecobonus e al sismabonus. Ricordo giornate infuocatissime, con agenzie di ogni tipo e colore.

per gli investimenti nel risanamento urbano e nella rigenerazione urbana e sostenibile. Si tratta di interventi importanti, basati su più annualità.

con riferimento ai contratti di filiera e distrettuali per i settori dell'agroalimentare, della pesca, dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo, a partire già da un primo importantissimo importo per il 2021 di 200 milioni di euro. Queste risorse - badate bene - sono aggiuntive rispetto agli 8 miliardi di euro già previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Pertanto, in totale parliamo di 9,2 miliardi certi, che creano un valore superiore a 25 miliardi nell'ambito di tutto l'agroalimentare, dalla terra alla tavola. Si tratta di misure straordinarie e importanti. Nell'ambito di questa strategia, e cioè l'agricoltura sostenibile e l'economia circolare, noi abbiamo portato avanti anche in 9a Commissione alcune indicazioni importanti che il Governo deve tenere presente nella definizione dei decreti attuativi: occorre accrescere la competitività del settore, investendo in formazione finalizzata alla diffusione dell'agricoltura 4.0, dell'agricoltura di precisione, all'utilizzo di molte tecnologie innovative connesse anche agli improvvisi e anomali cambiamenti climatici. Voi sapete che quest'anno il nostro Paese ha subito un danno da un miliardo di euro per le gelate. Noi dobbiamo prevenire, e non combattere, gli eventi con le risorse e questo diventa fondamentale e strategico per tutti i nostri agricoltori. dobbiamo promuovere un processo importante favorendo la rottamazione dei mezzi agricoli più vecchi, inquinanti e obsoleti, dando sicurezza, tranquillità e protezione al lavoro dei nostri agricoltori.

Dobbiamo altresì abbattere i costi di produzione e vi richiamo alla mozione presentata la scorsa settimana per quanto riguarda i costi delle materie prime. Dobbiamo intervenire per sburocratizzare le procedure, semplificare,

decreto semplificazioni, e ora dobbiamo aiutare l'imprenditoria femminile con risorse certe, contributi a fondo perduto e interessi in modo tale che possano investire nelle attività agricole. attuare una strategia importante a sostegno del *made in Italy,* sui canali sui quali si fonda l'antica tradizione culinaria del nostro Paese: la dieta mediterranea, straordinario elemento di propaganda nel mondo di quello è che il *made in Italy,* con certezza di salubrità del prodotto. Nella più famosa delle sue «Prediche inutili» Luigi Einaudi disse che il legislatore per deliberare doveva conoscere. Allora noi dobbiamo pensare che oggi il *brand* *made in Italy* nel mondo ha un valore di 1.700 miliardi di dollari; è diminuito rispetto agli anni scorsi, ma è sempre importante. Per questo dobbiamo agire secondo l'orientamento che noi diamo, perché tra i problemi più importanti, oltre quello della burocrazia e della cosa pubblica, c'è anche quello della giustizia. La Lega sarà quindi a fianco di tutti coloro che operano in questo settore con molta determinazione, per superare le criticità che ho citato poc'anzi e soprattutto per avviarci verso un percorso costruttivo e positivo per il nostro settore agroalimentare, vero pilastro del PIL. *(Applausi)*.

prima di chiarire alcuni aspetti tecnici contenuti nel decreto-legge relativo al Piano complementare oggi in esame, è necessario aprire velocemente un *focus* sui principali aspetti del contesto che ha reso necessaria l'emanazione di questo provvedimento economico, accanto a tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Già prima della pandemia l'Italia in Europa, o ancora meglio tutta l'Unione europea, era inserita in un perimetro di regole economico-finanziarie rigide, non al passo con le grandi sfide che i cambiamenti climatici e poi la pandemia ci avevano messo di fronte. La pandemia è stata un acceleratore dei processi di cambiamento ora più urgenti, avviati dalla netta

come anche a sospendere il Patto di stabilità e crescita e molte rigidità nelle regole sugli aiuti di Stato. La Banca centrale europea ha radicalmente cambiato la sua cassetta degli attrezzi, acquistando massicciamente titoli di Stato e dimostrando che non è certo un aumento del debito pubblico a incidere sul famoso *spread*, ma sono proprio le politiche monetarie della stessa BCE. Oggi ci troviamo a discutere e direi a raccogliere i frutti di tutto questo, seppur generati da un dramma umano e sociale qual è stato purtroppo la pandemia. Guardando al decreto-legge del Fondo complementare e, attraverso di esso, a tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il MoVimento 5 Stelle è riuscito a presidiare e garantire gli sviluppi di alcune misure fondamentali per il rilancio del Paese. All'interno del decreto, che - come sappiamo - stanzia 30 miliardi di euro da qui al 2026 per supportare progetti accanto al Piano nazionale, mi voglio concentrare su due misure targate MoVimento 5 Stelle, le più finanziate. Una riguarda

riguarda le agevolazioni negli investimenti per le imprese (transizione 4.0), a cui il decreto-legge assegna 5 miliardi, che salgono a oltre 18 miliardi, sempre come risorse complessive. La pandemia ha imposto la necessità di iniziare una corsa inarrestabile verso il futuro mettendo in campo strumenti rivoluzionari e processi completamente ripensati. E lo abbiamo fatto a partire dal decreto-legge rilancio con il superbonus 110 per cento sviluppando il meccanismo della cedibilità dei crediti di imposta. Su questo tema non può essere il parere ambiguo di Eurostat a condizionare il Governo a impedire che tale meccanismo venga esteso anche ai crediti d'imposta per gli investimenti delle imprese in transizione 4.0. Tutti gli osservatori economici individuano nella cedibilità del credito un fondamentale strumento per garantire l'immissione di liquidità a tutto il mondo delle imprese che ne ha necessità per superare le tante difficoltà e creare l'occupazione che serve. L'estensione di cedibilità del credito è stata anche sottoscritta, su *input* del MoVimento 5 Stelle, da tutte le forze politiche nella relazione finale del PNRR, e non può esserne impedita l'adozione proprio ora, mentre è in corso una profonda e inevitabile rivisitazione

per quanto riguarda me e il MoVimento 5 Stelle, sono convinta che con coraggio e determinazione lo stiamo facendo.

Credo che questo sia un buon provvedimento. Il decreto-legge del Governo, avendo le stesse finalità e le stesse linee guida del PNRR è un buon provvedimento e strutturato bene, con uno sguardo fisso verso il il futuro. E anche le misure adottate in Parlamento vanno nella stessa direzione e sono interessanti. Rassicuro anche i colleghi che sono preoccupati per le risorse al Sud: anche la Commissione bilancio ha lavorato per potenziare l'accessibilità e la sicurezza delle strade con particolare riferimento al Sud, alle aree interne, ai collegamenti di "ultimo miglio" con porti e aeroporti, ai Comuni di medie dimensioni e anche ai collegamenti con i siti archeologici. Non solo: è stato approvato un emendamento molto interessante che prevede una relazione annuale al Parlamento per monitorare la territorializzazione delle risorse, in modo che ciascun parlamentare possa tenere sotto monitoraggio questo percorso. Anche gli ordini del giorno presentati sono molto interessanti e importanti, perché il Governo ha accettato di impegnarsi affinché nei prossimi provvedimenti, a partire dalla legge di bilancio, possano possano essere messi in atto. Parlo - ad esempio - del potenziamento delle misure sui terremoti, quelli che in questo provvedimento sono rimasti esclusi, e della misura molto richiesta e importante del 110 per cento che permette la transizione *green* di tutti i nostri edifici, che noi conosciamo essere particolarmente datati. Anche un ampliamento soggettivo della misura del 110 per cento è importante in chiave di attività di impresa, proprio per sposare la visione di connubio tra capacità di fare impresa e di intraprendere in maniera sostenibile.

il debito che effettivamente nel suo rapporto con il PIL è arrivato quasi al 160 per cento. È quindi un debito buono che va nella giusta direzione. Finalmente, dopo 240 miliardi di indebitamento un po' passivo, andiamo nella direzione giusta. Sul percorso hanno ragione i colleghi:

perché è strettamente connesso e intrecciato al PNRR ed era di difficile emendabilità. Il fatto invece di esserci riusciti sia a livello ordinamentale, sia a livello di emendamenti onerosi, dà la prova di un grande lavoro e di collaborazione tra Governo e Parlamento.

Signor Presidente, vorrei ringraziare il Governo, il ministro D'Incà, i sottosegretari Bini e Sartore e, in particolare, il ministro Carfagna per la disponibilità a trovare spazi emendativi sul Fondo di sviluppo e coesione per 700 milioni.

sia nella fase emendativa, sia attraverso la trasformazione in ordine del giorno di temi significativi che ora sono all'attenzione del Governo per i prossimi emendamenti. Stiamo vivendo un momento storico che per difficoltà, per il debito che i giovani si sono accollati, per il non semplice rapporto, anche equilibrato, tra Governo e Parlamento, per la sfida che questa dotazione straordinaria di risorse ci impone, impone, speriamo possa permettere una fase di crescita espansiva e di progresso per le nostre imprese, per le nostre famiglie e per la parte più povera e sofferente del Paese, affinché possa esserci una reale e responsabile

Signor Presidente, cercherò di essere estremamente sintetico, visto che ci stiamo dando tempi molto limitati per le dichiarazioni di voto. Ci apprestiamo a votare un provvedimento che riveste un'importanza strategica

un miglioramento dovuto al lavoro fatto dalle Commissioni, che sicuramente vanno ringraziate in maniera molto sentita perché arrivare a una soluzione condivisa su temi così importanti non è cosa facile.

e lo devo dire - ci si dimentica che anche la Sardegna fa parte del Sud, che anch'essa fa parte del Mezzogiorno; è un'isola e quindi risente di tutte le

con la rapidità con cui ha operato in questa circostanza anche per trovare una soluzione efficace su altri fronti. In particolare, mi riferisco a una questione cruciale per l'intero Paese, ovvero la crisi della compagnia Air Italy, che sta sconvolgendo i trasporti nazionali e ancora una volta i trasporti fra la Penisola e la Sardegna. Mi auguro che entro brevissimo tempo il Governo si faccia carico di questo problema. So che oggi c'è stato un incontro - o forse è ancora in corso - tra i rappresentanti della compagnia e il Governo stesso.

corrono il rischio del licenziamento per una serie di motivazioni che non sono ancora completamente chiare; la cassa integrazione terminerà il 30 giugno. giugno. Visto che stiamo facendo operazioni tanto importanti, quali quelle previste da questo provvedimento che, come dicevo, integrano

Noi, come Gruppo Misto-LeU-Eco voteremo a favore di questo provvedimento. Sono state fatte alcune scelte importanti: la riqualificazione energetica nell'area adriatica per la produzione di energia rinnovabile, la digitalizzazione del sistema della scuola, i collegamenti ferroviari nel Sud, la riqualificazione urbana.

della pianura padana. Tuttavia si utilizza, costretti dalle condizioni oggettive, uno strumento (l'FSC) con un elemento complicato di procedura. Non potevamo fare diversamente per riconoscere un'impronta che giustamente tutti i Gruppi, compresa la stessa opposizione, hanno rivendicato. Voglio dire con chiarezza che spero che questo non rappresenti un precedente rispetto al tema dell'FSC, perché l'FSC non deve e non può più essere - su questo siamo tutti d'accordo - un bancomat che si utilizza a seconda delle necessità.

Ora, tutto questo si inserisce in uno sforzo straordinario di cambiamento del Paese; avremo modo di discuterne ancora. Noi abbiamo dato il nostro contributo nella discussione sul PNRR e pensiamo si debba avere la massima attenzione nella gestione in relazione non solo ai tempi dei progetti, ma anche alla loro qualità, a partire dalla corrispondenza in riferimento ai grandi obiettivi: transizione ecologica, donne, giovani, Mezzogiorno, lavoro. Queste sono priorità che vanno governate; avremo modo di discuterne con la semplificazione e con le scelte che il Governo dovrà fare. Visto che il tempo alla fine, vorrei porre con sincerità un problema più complessivo. In quest'Aula più volte abbiamo rivendicato il ruolo del Senato e del Parlamento. Diciamocelo, colleghi: è molto difficile realizzare questo impegno, ma è indispensabile. è indispensabile. Non possiamo - lo dico al Governo - procedere in una dinamica che sostanzialmente non consente un contributo reale del Parlamento, in questo caso del Senato. Intendiamoci, le ragioni per cui siamo qua sono note: la pandemia e l'emergenza, tutte ragioni più che fondate. A questo punto, chiediamo al Governo di farsi carico di questo problema non a parole, ma trovando un metodo che, pur nella dinamica dell'emergenza consenta ai Gruppi e al Parlamento di svolgere una funzione,

non rappresenta perché non svolge il suo ruolo, c'è un problema oggettivo per tutti, sia per il Paese che per la democrazia. Mi aspetto che il Governo

il vice ministro Castelli ha esordito dicendo - da subito - che il decreto era bloccato e che non vi erano le condizioni

per i nostri concittadini. E non ci siamo sbagliati, perché oggi ci troviamo in quest'Aula, dopo quasi un mese di incertezze, ad esaminare un provvedimento (che tra l'altro è molto snello perché formato da soli sei articoli), sul quale i partiti di Governo non hanno fatto altro che discutere e scontrarsi, mentre gli esponenti dell'Esecutivo, che in parte vedo presenti oggi, sono stati in vistoso imbarazzo e non hanno potuto far altro che bocciare molte richieste, in particolare le nostre, per mancanza di coperture finanziarie. Da settimane Fratelli d'Italia denuncia l'assenza di un vero e proprio dibattito sul Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, soprattutto nel metodo. Voglio ricordare che anche sul Piano nazionale di ripresa e resilienza il Parlamento ha di fatto perso mesi a discutere della bozza predisposta dal Governo Conte II, salvo poi ritrovarsi in Aula con delle comunicazioni del presidente Draghi e un provvedimento infiocchettato. Il Piano, preparato dal Governo, è stato vistato dalla Commissione europea addirittura prima che dal Parlamento nazionale. Le Camere non hanno potuto spostare neanche una virgola e hanno peraltro preso visione dei documenti completi in tutta fretta, visti i tempi stringenti dettati da Bruxelles. La conseguenza è che solo oggi veniamo a conoscenza di molti progetti nascosti tra le righe di questo Piano, come ad esempio

tramite un algoritmo che, collegato a diverse banche dati, avrà il compito di individuare comportamenti sospetti di potenziali evasori, con buona pace della *privacy.* Nel frattempo, siamo in attesa che il Piano nazionale di ripresa e resilienza divenga operativo. Sappiamo bene che tutto ciò non potrà accadere se non verranno varate le famose riforme; riforme corpose come quella della giustizia, della concorrenza e del Fisco, solo per citarne alcune.

sembrerebbe molto tempo, ma in realtà sarà molto poco. Senza queste riforme, come tutti sapete, sarà anche difficile portare avanti un piano così ambizioso, che deve trovare conferma entro il 2026. Signor Presidente, da quando siamo in emergenza forse qualcuno crede che si possa sospendere la democrazia, come si è tentato di fare in questi ultimi quindici prima a suon di *lockdown,* poi con provvedimenti ancora fortemente restrittivi della libertà personale, mentre nel frattempo si sospende anche il dibattito politico, lasciando agire come unico soggetto il Governo, peraltro neppure espressione di una volontà popolare. La verità è che in questi giorni forse siete stati troppo impegnati a scontrarvi in una maggioranza così variegata,

abbiamo anche sentito l'ex *premier* Conte elogiare ancora una volta il reddito di cittadinanza come misura di inclusione sociale da rivendicare con orgoglio; una misura - lo dobbiamo lo dobbiamo constatare con dispiacere - che è stata confermata e finanziata anche dal Governo Draghi, dal quale sinceramente ci saremmo aspettati ben altro. Forse solo a Fratelli d'Italia, perché gli altri sono sordi e muti, giungono informazioni su mafiosi, spacciatori, immigrati che percepiscono indebitamente il reddito di cittadinanza; milioni di euro sprecati che potevano essere destinati alle imprese per creare lavoro e che invece sono andati a sostenere persone sedute sul proprio divano di casa. Allo stesso modo è stato interessante sentire in questi giorni

siete troppo impegnati a cercare un modo per mettere le mani, come diceva il mio collega De Carlo, nelle tasche degli italiani a suon di patrimoniale o ad aprire i confini all'immigrazione clandestina, pensando che in questo momento agli italiani interessi lo *ius soli* piuttosto che la stabilità e la ripresa economica.

Tutto quello che non è entrato nel PNRR lo ha deciso l'Europa, non il Parlamento nazionale. Eppure non abbiamo chiesto la luna: abbiamo presentato appena quindici emendamenti, pochissimi, per dare dimostrazione, come sempre, che siamo un partito e un Gruppo responsabile che vuole il bene dei nostri concittadini. Noi a questo modo di fare e a questo confronto che c'è in maggioranza e non c'è nelle Aule del Parlamento non siamo disponibili, non ci piace e continueremo a denunciarlo. Ma, come abbiamo detto fin dall'inizio, il nostro stare all'opposizione di questo Governo sarà all'insegna della responsabilità e non della contrarietà a prescindere. Per questo, in nome della responsabilità che nutriamo nei confronti degli italiani e consapevoli delle aspettative contenute anche in questo provvedimento complementare al PNRR, con tutti i limiti che abbiamo rilevato, il voto di Fratelli d'Italia sarà di astensione. *(Applausi)*.

nel dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento, voglio solo limitarmi a due considerazioni,

anzi, il contrario: il Governo è più forte se salvaguarda la centralità del Parlamento nel pieno rispetto della Costituzione. Considero il lavoro svolto in questa conversione un primo segnale importante, perché siamo riusciti, grazie alla collaborazione sia all'interno della maggioranza ma soprattutto in relazione con il Governo, a dare un'identità al percorso della conversione. Stiamo infatti parlando di un provvedimento che completa il perimetro della programmazione europea,

Lo dico con affetto al collega Calandrini: ho sempre pieno rispetto delle prerogative delle opposizioni, però si può fare opposizione - lo dico soprattutto a Fratelli d'Italia - senza insultare il Governo e gli italiani. Il Governo in questa fase è impegnato in un'azione importantissima importantissima per gli italiani, cioè quella di restituire crescita e speranza, ridurre le disuguaglianze, dunque dare futuro al nostro Paese. Si può fare opposizione senza insultare gli italiani. Dunque, credo che questo importante provvedimento di conversione completi innanzitutto il perimetro dell'attuazione della strategia europea e del nuovo volto dell'Europa, che secondo noi non deve essere emergenziale, ma deve addirittura diventare strutturale per superare l'Europa dei vincoli e del Patto di stabilità, per costruire un'Europa della crescita e della conversione in chiave ecologica, dell'economia e della digitalizzazione del Paese. Ma soprattutto siamo di fronte a provvedimenti sugli investimenti di particolare rilevanza, dunque anche il lavoro che abbiamo svolto, ad esempio per impegnare una parte del Fondo per lo sviluppo e la coesione, lo considero prezioso, un primo impatto importante nell'esercizio della funzione centrale del Parlamento. Grazie alla disponibilità anche del ministro Carfagna, che voglio sottolineare, siamo riusciti ad indicare alcune priorità e alcuni progetti (700 milioni di euro) che sicuramente, pur nel rispetto delle prerogative e degli accordi di partenariato e del ruolo delle Regioni (che nessuno vuole far venir meno), indicano alcune grandi questioni centrali. Alcuni miei colleghi le hanno già richiamate, quindi per brevità ne cito solo alcune: ad esempio, l'importante progetto che riguarda la Pianura padana, per il contrasto all'inquinamento che ci porta sanzioni europee con costi enormi per il Paese

quindi contrastare e affrontare i temi di quest'area così importante per il Paese, per generare meno emissioni in atmosfera e avviare tale area verso processi *green*, di rigenerazione ambientale e energetica. secondo progetto importante che abbiamo sostenuto tutti insieme e che riguarda l'intervento nel bacino dell'Adriatico, soprattutto sul versante dell'eolico, dell'energia da fonti rinnovabili, della trasformazione di piattaforme verso una riconversione in chiave ecologica dell'economia. Credo che sia un segnale importantissimo dato da un Paese che abbraccia il futuro e respinge l'idea della resistenza e cioè dell'ambiente come vincolo alle fonti rinnovabili. Credo che tutto questo rappresenti rappresenti un segnale di grande attenzione sulle priorità del PNRR, che qualifica il Parlamento ed essere arrivati in Assemblea - penso per la prima volta - su un provvedimento economico così ampio senza il voto di fiducia,

infine al Governo il rispetto gli impegni presi negli ordini del giorno approvati dalle Commissioni perché ci sono importanti indicazioni del Parlamento che, in coerenza con la restituzione della centralità al Parlamento, devono essere adottate. *(Applausi)*. Ci sono questioni importanti che riguardano giovani donne, *bonus* energetico, superbonus e non solo, aree industriali da riqualificare;

La qualità della proposta politica, che tutti quanti noi stiamo enunciando in quest'Aula, è mostrata dall'emendamento da 700 milioni di euro

per ottenere provvedimenti che riguardano la rete di interconnessione nazionale dell'istruzione, la trasformazione di poli energetici *offshore* nell'Adriatico, la questione che riguarda una delle proposte di Forza Italia,

Un risultato assolutamente importante

con provvedimenti importanti, come quello in discussione, che cuba in totale oltre 30 miliardi di euro, che possono essere subito spesi

stiamo già facendo da molte settimane, perché ci stiamo impegnando su quella che deve essere la battaglia delle battaglie: la riforma fiscale che il Paese aspetta da anni e da tempo. *(Applausi)*. È una battaglia che invito tutto il Parlamento a fare al più presto, perché i cittadini ne hanno bisogno. Usciremo oggi da questa crisi soltanto consentendo alle nostre famiglie e alle nostre aziende di recuperare potere di acquisto e quindi, soprattutto, di rimettere in moto la nostra economia. È questa la sfida del futuro, è questa la sfida del nostro Paese.

lasciatemi innanzitutto ringraziare l'intera Commissione bilancio per il lavoro svolto, i colleghi, i funzionari e tutti gli uffici. Un ringraziamento particolare va al Governo

Questi momenti in 5a Commissione sono sempre duri, ma si riesce poi alla fine a trovare la quadra. Abbiamo tutti molte aspettative legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono risorse che arriveranno dall'Europa, a condizione che l'Italia sia in grado di attuare importanti riforme.

con l'ultimo scostamento (sono 30 miliardi aggiuntivi rispetto ai 191,5 miliardi attesi dall'Europa). Ovviamente dovremo saper essere veloci ed efficienti. Il lavoro parlamentare, come ho detto, è stato comunque faticoso, talvolta legato a complicate logiche di Gruppo, ma in realtà quello che occorre all'Italia è velocità, semplificazione e serietà da parte di tutti noi. È quello che abbiamo tentato di fare in Commissione bilancio in questi giorni. Gli emendamenti gli spunti di miglioramento sono stati condivisi dai Gruppi e recepiti e lavorati quindi con l'impegno forte del Governo. Voglio ricordare qui alcuni interventi su cui abbiamo potuto dare il nostro apporto, con argomenti importanti come la sicurezza stradale, la manutenzione dei ponti, le risorse per il turismo, per gli impianti eolici, per le energie rinnovabili a largo del mar Adriatico, per la qualità dell'aria nella Pianura padana. sono state accolte poi come ordini del giorno, che non devono rimanere lettera morta. In particolare, vorrei sottolineare l'importanza delle proposte sull'ecobonus del 110 per cento. Si tratta di una misura, di un'opportunità importante per rinnovare il patrimonio immobiliare dell'Italia, finalizzata all'efficientamento energetico nell'ottica della transizione ecologica. È importante, quindi, che il Governo colga gli spunti proposti dal nostro Gruppo perché la misura sia prorogata al 2023, misura già annunciata per la prossima legge di bilancio, ma qui rafforzata e richiesta nei nostri emendamenti trasformati in ordine del giorno, perché è assolutamente importante dare sicurezza agli operatori del settore e a coloro che intendono avvalersi di questa misura. Con riguardo alla questione dell'attivazione dei provvedimenti, abbiamo anche elaborato alcune proposte volte ad ovviare al problema dei costi delle materie prime. Questo è un tema che personalmente tengo sotto osservazione da inizio anno, di cui il Governo deve avere contezza. Abbiamo quindi bisogno di realizzare i progetti, ma a causa della carenza delle materie prime e del conseguente aumento dei prezzi, si rischia il blocco dei lavori e si rischia che alcuni importanti interventi già programmati

a questo problema particolare. Colleghi, questo fondo complementare deve servire, come dice il nome, a completamento dei fondi previsti per il *recovery plan*, a riuscire a finanziare il disegno complessivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma tengo ancora a ricordare che a fronte di questo fondo, che è debito pubblico di immediata emissione, i 191,5 miliardi attesi dall'Europa sono condizionati, quindi dovremo essere veloci ed efficienti e questo è l'impegno che tutti noi

una dotazione di 30 miliardi, risorse che saranno utilizzate nell'economia reale per gli investimenti e per costruire un futuro più equo e più sostenibile. Come dice la sua stessa intitolazione, è un fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e di resilienza che ad oggi per l'Italia ammonta a complessivi 235 miliardi fino al 2026. al 2026. Tengo e teniamo a sottolineare e a ribadire che senza l'impegno profuso in Europa dal Governo Conte II e dal suo presidente del consiglio Giuseppe Conte, che noi abbiamo appoggiato convintamente e lealmente per tutta la durata del suo mandato, questo risultato non sarebbe non sarebbe mai stato conseguito e quindi ne siamo particolarmente orgogliosi. La misura contiene molti interventi davvero importanti, viene finanziato ulteriormente il superbonus

ambiamo a che questa misura venga ulteriormente prorogata, perché ha dimostrato i suoi effetti sull'economia reale e quindi, dal nostro punto di vista, dovremmo approvare il prima possibile questa proroga, magari non aspettando la legge di bilancio. Ulteriori finanziamenti sono stati destinati al piano Transizione 4.0, che è stato finanziato ulteriormente per 5 miliardi. Sono inoltre previsti interventi infrastrutturali, ad esempio sull'alta velocità, sulla Salerno-Reggio Calabria; è stato rifinanziato il fondo per lo sviluppo e la coesione per 15,5 miliardi e sono stanziati nuovi fondi per il terremoto

la cedibilità dei crediti fiscali per quanto riguarda la Transizione 4.0. È una norma che riteniamo davvero fondamentale per dare respiro e liquidità alle imprese e per arrivare a quello che abbiamo soprannominato il superbonus imprese. Lo chiede praticamente tutto l'arco parlamentare, che si è accodato - e noi ne siamo felicissimi - alla battaglia e alla richiesta del MoVimento 5 Stelle, ma soprattutto ce lo chiedono tutte le principali associazioni di impresa come Confindustria, Confagricoltura, la CIA, Confapi, Copagri, ABI e Coldiretti solo per citarne alcuni. Noi, in qualità di convinti proponenti di questa misura, ci batteremo finché diventerà norma dello Stato e non sarà certo per Eurostat o per il parere di un burocrate europeo, i cui peraltro rispettabili dubbi provengono però, forse, da chi non ha ancora capito che il mondo postpandemia è cambiato per sempre e non ritornerà più lo stesso. Non sarà certo questo parere a fermarci o a fermare un intero Paese, che ha solo voglia di lavorare, di riacquisire fiducia, di risollevarsi, di tornare grande e di progettare un futuro migliore, più equo e più inclusivo. Dobbiamo proseguire sulla strada del coraggio e dell'innovazione, sia nel campo economico e finanziario, sia in quello politico. Lo dobbiamo ai cittadini, lo dobbiamo a un'intera società che ha sofferto in modo incredibile in questi ultimi lunghi mesi di pandemia. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge da parte del MoVimento 5 Stelle.

è che, nel sottinteso di tutti questi provvedimenti, ogni tanto si infila la manina diabolica di qualcuno, che va a cancellare i sogni delle riprese. Nel PNRR, a pagina 58, ci sono due righe che da sole costituiscono una bomba sociale annunciata. Infatti a pagina 58 è scritto che: «si abrogano le disposizioni del codice di procedura civile» e le leggi che si riferiscono alla formula esecutiva. Tra l'altro questo è un cambio di passo rispetto al progetto precedente, in cui si scriveva: «si propone di abrogare»; invece, a pagina 58 del PNRR, si dà già la licenza di abrogare. Questa mi sembra tanto una scrittura ispirata dal sistema bancario, che rischia non soltanto sotto minaccia le famiglie sottoposte ad asta immobiliare, ma anche, ancora una volta, di farci tornare a una situazione cui, con il primo Governo, avevamo in qualche modo rimediato con la famosa legge Bramini. Non capisco quindi lo spirito di questa riforma del codice di procedura civile, in nome della velocità. Mi sembra che tutto sia ispirato da un sistema bancario. Vedo che adesso qualcuno ha capito che coloro che manterranno la sospensione delle rate rischiano una riclassificazione a *forborne* che, di fatto, è un primo *step* prima della segnalazione alla centrale rischi per essere inclusi nella categoria del credito problematico.

tutte le parole di fiducia e di speranza, però stiamo attenti, perché stiamo costruendo un edificio in cui l'economia reale e le famiglie rischiano di essere minacciate dal sistema bancario e finanziario.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della cultura, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

nell'interrogazione che abbiamo presentato come Gruppo Italia Viva-PSI vogliamo porre l'attenzione su uno dei settori che è stato più duramente colpito dall'emergenza Covid, in modo particolare la cultura e il turismo. Non serve ricordare in questa sede l'importanza strategica di questi due settori. Basti solo pensare - per avere un'idea - che il il turismo assume un valore di circa il 12 del PIL nazionale. Sappiamo che tra i settori nevralgici su cui punta il PNRR vi sono proprio la cultura e il turismo. sappiamo che sono previsti investimenti di quasi 7 miliardi di euro, finalizzati anche a incrementare il livello di attrattività di questi comparti attraverso la modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali, così come è previsto uno stanziamento di 300 milioni di euro a favore di interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive. Un simile intervento va sicuramente nella direzione giusta, ma pensiamo che non sia ancora del tutto sufficiente, guardando solo ai numeri - ad esempio - delle persone disabili in Italia, che sono più di tre milioni. Riteniamo Riteniamo quindi - ecco il senso dell'interrogazione che abbiamo proposto - che sia necessario intervenire in maniera ancora più incisiva, estesa e diffusa a favore della rimozione delle barriere architettoniche nei luoghi di fruizione della cultura e del turismo. tempo pensiamo sia necessario prevedere interventi di sostegno e promozione dei lavoratori dello spettacolo, al fine di ristorare e tutelare questo comparto che non ha trovato ancora un riconoscimento adeguato nel PNRR. Auspichiamo Auspichiamo che - anche dalla risposta che oggi ci darà il Ministro - si possa essere ancora più propositivi verso un settore davvero importante per la ripresa del nostro Paese.

in sede di predisposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, proprio per consentire un accesso più ampio dei cittadini nei luoghi della cultura, il Ministero ha previsto uno stanziamento di 300.000 milioni di euro volti al superamento delle barriere architettoniche senso-percettive, culturali e cognitive, e al rafforzamento delle competenze degli operatori. La presenza delle barriere architettoniche costituisce infatti ancora una criticità molto forte nei luoghi della cultura italiana, come è stato evidenziato dal rapporto annuale sui musei dell'Istat del dicembre 2019. Solo il 53 per cento di musei, monumenti, aree archeologiche e parchi statali e non statali ha migliorato le proprie strutture, rimuovendo le barriere fisiche; solo il 12 per cento ha superato le criticità collegate alle barriere percettive, culturali e cognitive. L'investimento del PNRR è quindi rivolto prioritariamente ai siti culturali statali dislocati su tutto il territorio nazionale, mentre una quota, che si potrà discutere stiamo discutendo di questo proprio con le Regioni - che nelle indicazioni della scheda è pari al 10 per cento, ma potrà aumentare, è destinata a musei regionali, provinciali e civici, gestiti da enti pubblici da organizzazioni senza scopo di lucro. Anche attraverso tale intervento si prevede di poter conseguire il superamento delle barriere architettoniche nell'80 per cento dei musei, aree e parchi archeologici e delle barriere senso-percettive nel 50 per cento delle medesime strutture. Questo concorre ovviamente al superamento delle diseguaglianze e dei divari che impediscono a tutti i cittadini di partecipare pienamente alla vita culturale del proprio territorio. In questo senso raccolgo molto volentieri l'invito della senatrice interrogante, volto a sostenere, attraverso nuove misure, l'abbattimento delle barriere anche in altri luoghi della cultura diversi dai musei. Ci lavoreremo sia con le risorse previste da PNRR che con le risorse ordinarie, perché naturalmente l'esigenza di questo tipo di intervento non finisce con l'utilizzo delle risorse del PNRR. Inoltre, relativamente al sostegno alle bande musicali e alla musica, ricordo che i decreti ministeriali 2020-2021 hanno riconosciuto ristori in loro favore, considerando ammissibili, tra gli altri, anche i costi sostenuti per l'acquisto di materiali e strumenti musicali, oltre che di spartiti, leggii e divise. Quindi è una novità su cui continueremo a lavorare, perché si tratta di un settore che merita assolutamente il più ampio riconoscimento.

So quanto lei sta lavorando in tale direzione. Auspichiamo che, anche attraverso questa sollecitazione ulteriore, si possa migliorare il livello di accessibilità ai luoghi della cultura e del turismo - come lei ha giustamente appena evidenziato - inclusi anche investimenti in strumenti musicali e misure di sostegno e promozione per i lavoratori dello spettacolo dal vivo, al fine proprio di tutelare questo comparto, che - come dicevo all'inizio - non ha trovato ancora un adeguato riconoscimento nel PNRR. Senza alcuna pretesa di esaustività, vorrei dedicare pochi minuti a questo importante comparto, stiamo inaugurando una pagina diversa con le riaperture; finalmente si potrà avere un po' di sollievo per le persone che hanno veramente sofferto moltissimo. In questi giorni riaprono teatri, musei e cinema. Auspichiamo, quindi, che a breve possano essere date indicazioni ancora più precise riguardo alle capienze. Finisco col dire, attraverso un libro che è appena uscito («Lucean le stelle» di Stefania Sandrelli e Alberto Veronesi),

Signor Ministro, il 31 maggio abbiamo registrato l'esordio della piattaforma digitale Itsart, da lei fortemente voluta: un progetto ambizioso, largamente condivisibile, che si prefigge di divulgare e rappresentare la cultura italiana in Italia e soprattutto nel mondo; un progetto che una Nazione come l'Italia deve avere e che onestamente ha trovato in noi anche delle convergenze (assolutamente sì). Certo, ci saremmo aspettati un nome più evocativo, un nome che tenesse conto della tradizione millenaria dell'Italia e non il solito copia-incolla, il solito tributo da pagare al politicamente corretto e al provincialismo esterofilo del quale purtroppo troppo spesso la nostra Nazione tende in qualche modo a vestirsi. Ma non è solo questo il problema; questo è l'ultimo dei problemi. Il problema più grande è invece quello che viene certificato come un vero e proprio fallimento di questo suo progetto. non lo dico io, ma lo dicono i giornali amici del suo partito; lo dicono tutti coloro che si aspettavano qualcosa di più a livello sia comunicativo che sostanziale. La mia domanda è la seguente: i circa 20 milioni di euro di soldi pubblici che il Ministero della cultura e Cassa depositi e prestiti hanno investito nel progetto non potevano essere usati forse per potenziare Raiplay oppure essere destinati agli operatori del mondo dello spettacolo che da quasi due anni non percepiscono un euro? Ministro, su questo vorrei una risposta.

sono andate spontaneamente sui siti delle varie istituzioni culturali e dei teatri, avendo un allargamento di pubblico molto forte che ha sostituito temporaneamente la presenza in sala. Su questo si sono innestate anche negli ultimi mesi delle esperienze all'estero di eventi che si sono spostati direttamente *live*, ma *online*. La scelta nasceva dall'idea di colmare provvisoriamente e transitoriamente la fase sia della chiusura che delle riaperture parziali con le limitazioni numeriche che ancora oggi caratterizzano l'apertura dei teatri e dei cinema; e ciò anche per avere un luogo che possa offrire all'Italia, agli italiani e a tutto il mondo gli spettacoli e gli eventi dal vivo che si svolgono in Italia di vario tipo (musica, teatro, danza e cinema),

acquistando i biglietti a un prezzo inferiore, partecipare a quell'evento, cosa che La Scala ha già anticipato con eventi nelle sale cinematografiche in diretta negli anni passati. È uno strumento tecnologicamente possibile. Da quel momento in poi, come prevedeva la norma, la gestione è stata affidata a Cassa depositi e prestiti, che ha scelto il *partner* privato e il nome. Ha fatto tutto autonomamente ed è giusto che la politica non interferisca né nella scelta dei contenuti, né negli strumenti a disposizione. Perché parlare di fallimento? Capisco che ci sono il dibattito politico e una certa fretta della stampa, ma parlare di fallimento e di *flop* - come ho letto - una settimana dopo la partenza è veramente un po' strano. È chiaro che è un meccanismo che andrà a crescere. I numeri che la società mi ha fornito al momento sono i seguenti: 400.000 accessi alla piattaforma, 35.000 utenti registrati, 120 *streaming* sui contenuti in catalogo che sono più di 700. Naturalmente è una piattaforma che deve crescere, l'invito a tutte le istituzioni culturali è offrire e mettere sulla piattaforma in vendita per avere delle entrate per i loro bilanci, aiutando contemporaneamente gli enti e offrendo un luogo in cui in Italia e dall'estero ci sarà la possibilità di accedere ai contenuti dell'offerta culturale italiana. Io inviterei - non mi preoccupo più di tanto, perché sono stato anche io all'opposizione - ad aspettare prima di parlare di *flop*. È un meccanismo che sta crescendo settimana dopo settimana; crescono i numeri dei contenuti inseriti

Non vorrei essere omissivo. Dall'inizio si è cercato di coinvolgere la RAI. Abbiamo ragionato di questo anche in Commissione vigilanza. In queste ore sono in corso contatti tra la RAI e la società che gestisce la piattaforma Itsart per creare forme di collaborazione che la RAI stessa ha ritenuto autonomamente non gestibili in quella forma, perché vende solo contenuti propri e non prodotti da altri.

registra teatri vuoti e spettacoli di piazza che non possono essere svolti. Magari ci si sarebbe aspettato, visto che parliamo anche di soldi pubblici, un intervento diverso.

il Lombroso è definito il padre della psicologia criminale, nonostante la scienza (non solo postuma, ma anche a lui contemporanea) abbia dichiarato infondate tutte le sue teorie, definendole pseudoscientifiche. Andrea Verga lo sconfessò miseramente sulla celebre fossetta occipitale su cui Lombroso fondò le sue teorie. Egli non gli rispose mai, tanto che per questo fu cacciato dalla Società di antropologia nel 1882. La convinzione di Lombroso si basava in particolare sulla tesi dell'uomo delinquente, nato atavico; insomma, il delinquente per natura, individuo che recherebbe nella struttura fisica i caratteri degenerativi che lo differenziano dall'uomo normale. Cito solo due brani di Lombroso per far capire quali fossero le sue idee sui meridionali: «Il meridionale non ama i liquori: si sente ebbro dalla nascita: il sole, il vento, gli distillano un terribile alcool naturale, di cui tutti quelli che nascono là giù ne sentono gli effetti». A proposito delle Regioni meridionali d'Italia, ebbe a dire: «La debolezza dell'Italia è nelle ginocchia, è alle gambe, ai piedi; il male, il male vero profondo è qui». Invito a considerare quanto segue. L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. distinte. A Torino ha sede il museo di antropologia criminale dedicato a Lombroso, che teorizzava - appunto - la presenza di due razze; sul sito del museo si legge che il nuovo allestimento vuole fornire al visitatore strumenti concettuali per comprendere come e perché questo personaggio così controverso formulò la teoria dell'atavismo criminale. Il museo è stato concepito con una funzione educativa intesa a mostrare come la costruzione della conoscenza scientifica sia un processo che avanza grazie alla dimostrazione non tanto di verità, quanto della falsificabilità di dati e teorie che non resistono a una critica. A tutt'oggi il museo non sembra assolvere alla sua funzione e veicola un messaggio sbagliato su cosa sia scienza. Quelli di Lombroso furono non errori scientifici, ma vere e proprie manipolazioni pseudoscientifiche fatte in malafede per interessi estranei alla scienza e le sue teorie furono funzionali a una propaganda di potere. Di questo il museo non rende conto. Vi ho fatto visita, insieme a una delegazione,

criminologo e antropologo Cesare Lombroso dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi del Novecento. Si tratta di collezioni eterogenee composte da crani, scheletri, disegni, corpi di reato, produzioni artigianali, eccetera. Dopo diversi sedi, nel 2001 è ospitato nel Palazzo degli istituti anatomici nell'ambito del polo dedicato al positivismo scientifico torinese. Lombroso è conosciuto per le sue teorie nel contesto della scienza positivista e il suo lavoro, sebbene oggi giustamente respinto dagli studiosi, costituisce un pezzo dello sviluppo dell'antropologia fisica. Il museo intende spiegare il processo che portò Lombroso allo sviluppo delle sue teorie nell'ambito dell'atavismo criminale, evidenziando l'infondatezza dei suoi metodi scientifici. L'allestimento odierno ha come obiettivo non quello che aveva all'origine, ma tutt'altro, ossia far conoscere il pensiero di Lombroso calato nel periodo in cui visse, spiegando le ragioni storiche e culturali e dimostrando l'assoluta infondatezza del pregiudizio fisiognomico - da un lato - e - dall'altro - come la scienza proceda proprio attraverso errori e correzioni. Il ruolo che il museo si propone è dunque quello di spiegare al pubblico una parte controversa del pensiero scientifico, che peraltro collide inevitabilmente con l'attuale sensibilità sociale, preservando la memoria in modo critico. Ricordo infine che la commissione etica dell'Organizzazione internazionale dei musei (ICOM), interpellata dal Comitato no Lombroso, ha rivisto già in passato tutti i documenti che riguardano il museo di antropologia criminale, condividendo la porzione di ICOM Italia che ha sottolineato come il museo rispetti gli *standard* scientifici e didattici per rimanere aperto. Pertanto, la risposta sulla chiusura è negativa. Anche se volessi, io non posso chiudere il museo. Ma, se potessi, non lo farei perché il mio compito è aprire musei e non chiuderli.

in cui il processo della memoria non venga sottoposto ai canoni della verità scientifica e anche storica. Tutte le inesattezze compiute da questo pseudoscienziato non sono facilmente ricavabili da una visita al museo, che nell'immaginario collettivo trasmette ancora l'idea l'idea di inferiorità razziale per le popolazioni meridionali che non meritano un simile trattamento. Soprattutto, riguardo al metodo scientifico, di cui pure c'è menzione in qualche pannello, che esso non consiste solo nello sbagliare e correggersi, ma nello sbagliare e correggersi pur avendo applicato i canoni della logica sperimentale. Noi siamo quindi di fronte a una persona che gli scienziati avevamo già definito non essere uno scienziato,

e potrebbe essere valorizzato, piuttosto che continuare a tenere in vita un museo che è l'equivalente di Mengele e si noti che ad Auschwitz non c'è un museo su Mengele.

al pari della musica lirica, il balletto classico è una delle principali ragioni la popolarità dell'Italia nel mondo. Noi abbiamo inventato entrambe le forme di espressione artistica e le abbiamo onorate nel tempo, offrendo ai palcoscenici del pianeta i migliori talenti internazionali, sia nel melodramma sia nel balletto classico. E questo ci giova, perché ha contribuito ad alimentare e a migliorare la reputazione internazionale dell'Italia in una fase storica in cui la reputazione è quasi tutto - credo sinceramente - contribuendo anche a far leva sul turismo e sull'*export.* signor Ministro, abbiamo un problema: delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche del Paese, soltanto quattro hanno mantenuto i loro corpi di ballo; le altre dieci li hanno dovuti dismettere, e non certo per ragioni artistiche, ma per evidenti questioni di bilancio per abbattere i costi. Esistono però dei costi immateriali che sono lievitati di conseguenza e che vengono pagati quotidianamente dai migliori artisti, dai migliori talenti della danza italiana, costretti

Tutto questo è ancor più paradossale tenendo conto che mai come oggi la danza, il ballo sono popolari. Credo che buona parte del merito vada attribuito ai *talent show* televisivi, e allora ben vengano anche loro. Abbiamo circa 30.000 scuole di danza in Italia che coinvolgono dai due i tre milioni di ragazzi. Questa è un'attività che va sostenuta concretamente e fiscalmente; va favorita perché incoraggia nei più giovani quelle virtù che lo spirito dei tempi inevitabilmente scoraggia e, quindi, l'attività fisica, la regola il senso del dovere, l'etica del sacrificio, la grazia. Pertanto, signor Ministro, Forza Italia le chiede davvero con forza di mettere il ripristino dei corpi di ballo nelle fondazioni lirico-sinfoniche al centro dell'azione riformatrice nel settore dello spettacolo e di conseguenza di ripristinare o quanto meno di incoraggiare quelli che un tempo chiamavamo enti lirici a riappropriarsi delle proprie funzioni istituzionali sin dal nome, denominando di conseguenza le fondazioni in liriche, sinfoniche e di balletto.

Come sapete, siamo intervenuti sui lavoratori dello spettacolo sia con misure d'urgenza nel decreto-legge sostegni, sia con misure - che avevamo annunciato - di recepimento dell'indicazione di un disegno di legge collegato materia di spettacolo, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri e che ora arriverà in Parlamento per l'approvazione. Quella è la sede propria in cui i parlamentari potranno fare queste riflessioni unitamente al Governo, e il Governo le sosterrà. In particolare, con specifico riferimento ai corpi di ballo, ricordo che la normativa in materia, attribuendo alle fondazioni lirico-sinfoniche la produzione di spettacolo e anche di balletto, non richiede che questi si avvalgano obbligatoriamente di un proprio corpo di ballo. Questo è rimesso pertanto alla valutazione degli amministratori che, con la crisi con la crisi economico-finanziaria che ha portato negli ultimi anni al commissariamento di ben dieci teatri e al confronto con le organizzazioni sindacali, devono valutare singolarmente l'opportunità di istituire nuovi corpi di ballo. In questo senso, nel mese di febbraio scorso, a seguito dell'adozione del decreto interministeriale che prevede lo schema tipo di dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche, ciascuna fondazione è stata invitata a formulare una proposta di dotazione organica da trasmettere ai Ministeri vigilanti, previa delibera del consiglio d'indirizzo (ovviamente sentiti i sindacati e le organizzazioni). Tale proposta deve essere corredata da un'apposita documentazione che attesti la sostenibilità economico-finanziaria, adeguati livelli di produzione di proprietà e numero di contratti di lavoro a tempo determinato riguardanti un biennio. È evidente che, in questo quadro che deve rispettare delle compatibilità finanziarie, c'è uno spazio

- è un po' difficile stabilire l'obbligatorietà del corpo di ballo -, prevedano degli incentivi o dei sostegni alle fondazioni lirico-sinfoniche, e queste ultime faranno la scelta di mantenere un corpo di ballo all'interno delle proprie attività. Siamo dunque prontissimi a lavorare

ad esempio ripartendo adeguatamente e integrando i fondi del FUS, affinché tutte o quasi le fondazioni lirico-sinfoniche siano incentivate a dotarsi dei corpi di ballo, che un tempo avevano e che ormai

amministrazione, e mettere noi parlamentari in grado di capire e di chiarire una questione per noi strategica come quella riguardante le assunzioni nella pubblica amministrazione. Si inaugura un periodo di riforme strutturali soprattutto con il PNRR e per il PNRR, che noi ci auguriamo faccia fare un salto di qualità, ormai atteso da anni, alla macchina statale. Questa è per noi un'opportunità strategica che siamo convinti il Governo abbia colto immediatamente anche in questo senso. Avere una pubblica amministrazione rinnovata ed efficiente è fondamentale per vincere anche la sfida del PNRR nella gestione di quelle risorse importanti che poi dovranno essere dispiegate nei territori. Noi, infatti, plaudiamo al Governo che ha subito scelto di spendersi in questo senso anche con

2.800 profili per irrobustire la capacità amministrativa di diversi enti locali e territoriali delle Regioni del Sud, anche al fine di gestire al meglio i progetti europei. Hanno partecipato in moltissimi. Più di 81.000 persone hanno presentato la domanda, avendone i requisiti; 8.000 e più sono stati gli ammessi, anche se purtroppo soltanto un terzo di questi si è presentato

l'immissione di questi profili professionali specialistici, perché queste erano le indicazioni della legge di bilancio per il 2021, al fine di dare specialisti, soprattutto in fondi comunitari, alle amministrazioni del Sud.

con un risultato da valutare relativamente basso. Quello che abbiamo fatto, proprio per onorare i 2.800

per un'area speciale come il Sud, cosa di solito non prevista dai concorsi pubblici, dedicato al Sud per ragioni ovviamente comprensibili. Per quanto riguarda poi i giovani, non c'entra assolutamente niente,

rispetto a concorsi con profili *standard* senza esigenze particolari, ma nel contempo anche le professionalità. Dovremo fare un salto di qualità che è previsto in Europa, per cui anche contratti a termine possano essere appetibili per professionisti qualificati, proprio per fare un'esperienza adeguata nella pubblica amministrazione. Resto comunque a vostra disposizione per spiegare questa rivoluzione che è in corso,

che la necessità prioritaria è quella di non perderle; perché ciò non accada, abbiamo bisogno di enti locali forti, che abbiano strutture in grado di lavorare soprattutto sui progetti europei.

*(M5S)*. Egregio Ministro per la pubblica amministrazione, si è recentemente svolta la prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 2.800 tecnici per le amministrazioni pubbliche delle Regioni del Sud, bandito ai sensi del decreto-legge n. 44 del 2021. La procedura concorsuale prevista nel bando si articola in due fasi: la preselezione per titoli ed esperienza professionale, distinta per i diversi profili del concorso finalizzata all'ammissione alla prova scritta, e la seconda fase, che prevede una sola prova scritta selettiva, anche se distinta per i diversi profili. Questa nuova tipologia di procedura concorsuale, che prevede la preselezione in ingresso tramite valutazione dei titoli e delle esperienze professionali possedute dal candidato, è stata fortemente criticata soprattutto dal MoVimento 5 Stelle in fase di esame parlamentare del provvedimento e conseguentemente modificata nel testo del decreto convertito in legge, per quanto riguarda le prossime procedure concorsuali da realizzare. Non è stato però possibile attuare tale modifica ai concorsi già banditi, come quello in oggetto. Tale modalità di reclutamento ha quindi sicuramente penalizzato i giovani neolaureati e con meno possibilità economiche rispetto a coloro che sono in possesso di più titoli di studio e professionali. Il concorso ha visto un'elevata mancata partecipazione alla prova scritta e ciò ha indotto il dipartimento della funzione pubblica, nell'assoluta necessità di garantire l'interesse pubblico di vedere ricoperte tutte le le 2.800 posizioni ricercate, ad annullare la soglia di sbarramento per la partecipazione alla prova scritta e ad ammettere gli altri 70.000 candidati, ossia il 90 per cento di quelli che avevano presentato la domanda, che erano già stati scartati nella fase preselettiva. scelta, in conclusione, la linea dell'eliminazione della fase preselettiva per titoli, la stessa sostenuta dal nostro Gruppo e che era stata adottata in sede di conversione del decreto-legge. sono stati comunque esclusi dal concorso coloro che non avevano presentato la domanda, scoraggiati esclusivamente dalle nuove regole, perché consapevoli di non poter contare su una formazione specialistica ed esperienze professionali pregresse. Pertanto le chiedo, signor Ministro, quale sia la valutazione di questi fatti; quale sia, per ogni profilo bandito, il numero delle richieste pervenute e il numero delle persone che si sono effettivamente presentate per sostenere la relativa prova scritta; se non ritenga che i requisiti di preselezione previsti nel bando siano stati non correttamente proporzionati rispetto ai profili banditi; se non ritenga che i profili banditi non siano stati inquadrati in un livello retributivo adeguato a tali funzioni e che ciò abbia determinato l'alto tasso di rinuncia alla partecipazione alla prova scritta.

com'era. Era un concorso speciale, per profili speciali, per dotare gli enti locali del Sud di professionalità speciali. Richiedeva quindi profili speciali, non per per neolaureati anche con lauree triennali (come prevede la legge), ma per persone con esperienza e con specialità di competenze. Questa era la natura di quel concorso.

le specializzazioni (perché, se il posto messo a concorso è *standard*, non richiede specializzazioni particolari), e profili (ed è stato un emendamento proprio del Senato a prevederlo) con caratteristiche di specialità tecnica, per i quali invece, ovviamente, è necessaria una valutazione dei titoli, come nel caso del concorso Sud. Pertanto, ciò che è stato fatto,

il decreto reclutamento che arriverà in quest'Aula la prossima settimana, anche far scorrere ulteriormente la graduatoria, partendo da questo concorso, al fine di dotare le amministrazioni del Sud di questi particolari profili. Il punto nodale, su cui abbiamo tanto discusso e che mi piacerebbe ancora di più discutere, è il seguente: contemperare l'esigenza dei giovani di avere un percorso e un ascensore sociale dai concorsi pubblici con quella di chi, non essendo più giovanissimo o neolaureato, ha però acquisito titoli legali, legalmente riconosciuti, di professionalità, che dovrebbero valere nei confronti di bandi speciali per posti speciali. Dovremmo tenerne conto e l'articolo 10 del decreto-legge n. del 2021 lo fa. Ad esempio, a Roma si sta svolgendo un concorso per dirigenti, ma anche per profili *standard*, che applica le due caratteristiche. Pertanto,

quando saremo a regime, fuori dalla pandemia, con un'eventuale prova orale; con la duplice valutazione, dei titoli legalmente riconosciuti, che serva di preselezione, ovvero con nessuna valutazione, se il tipo di posto messo a concorso è di carattere *standard* o generale. Questo consente di tener conto delle due esigenze: quelle di chi ha investito in formazione e quelle di chi non ha ancora potuto farlo, perché è giovane. Quindi, contemperiamo le due istanze, dando i segnali giusti: non perdere tempo con formazione mnemonica su quiz preselettivi imparati a memoria, ma investire su se stessi, stante la rigorosità delle prove concorsuali. Questo concorso Sud è l'ultimo di una serie, forse il primo di un'altra, e sarà bene riflettere tutti sul perché,

in funzione del PNRR, quando cercheremo decine di migliaia di professionalità specifiche, che temo non troveremo. Bisognerà fare una riflessione tutti insieme, su come reclutare e valutare, tenendo insieme qualità, ma anche necessità di capitale umano per i nostri enti locali. Questo è un problema che riguarda tutti. Siamo in una transizione da un vecchio sistema a uno nuovo e c'è bisogno dell'intelligenza collettiva di tutti noi, ossia del Parlamento, che è l'unico luogo dove tali questioni si possono e si devono discutere, proprio per rispondere alle esigenze straordinarie e strategiche del nostro Paese. Quindi, vi ringrazio sentitamente per questa piccola sessione di riflessione. Avremo modo di discuterne

Signor Ministro, la ringrazio per la risposta. Sono d'accordo con lei sul fatto che la pubblica amministrazione compiuto un passo nel rinnovamento dei concorsi. Quindi, sono anche d'accordo sulle strade intraprese in merito alla digitalizzazione e alle semplificazioni procedurali, che permettono di reclutare di offrire la risposta alla domanda di reclutamento in un tempo veramente più breve. Questa è una delle istanze che appunto anche i giovani che abbiamo incontrato e che ci hanno interpellato hanno posto. Una delle questioni è appunto quella fare la domanda al concorso e ricevere velocemente la risposta. La questione della scarsa appetibilità della pubblica amministrazione è una domanda che ci dobbiamo fare. È proprio questa la domanda contenuta nell'interrogazione, proprio perché, appunto, se richiediamo profili speciali, dobbiamo dare anche retribuzioni speciali, e questo non si è verificato con il concorso, in quanto quanto probabilmente i candidati, al momento della presentazione della domanda, non erano consapevoli del livello di retribuzione. ha esperienze e titoli professionali da far valere, si aspetta anche che magari il livello di inquadramento possa essere superiore. Auspichiamo che ci sia questa riflessione che permetta di contemperare due esigenze: da perché abbiamo bisogno anche di giovani che possano entrare da neolaureati, ricevere un percorso di formazione professionale

2021, ha introdotto, all'articolo 114, il riferimento alla città di Roma come capitale della Repubblica.

capitale degna di quest'Europa pari a Berlino, Madrid, Vienna o Bruxelles, anzi, Washington - ci allarghiamo con gli esempi - perché è la capitale della cultura non solo europea, ma anche mondiale. 6.000 chilometri di siti archeologici che devono essere gestiti in maniera costruttiva, indipendente, anche per dar seguito a tremila anni di storia. Per questo le chiediamo, signor Ministro, quali siano le indicazioni del Governo per arrivare

È questa la nostra domanda: cosa sta facendo il Governo per far diventare Roma, una volta per tutte, la capitale più importante d'Europa?

poteri e funzioni adeguati al ruolo che questa città ricopre, ma anche alla complessità dei problemi e alla vastità del patrimonio dell'Urbe, ricordando la configurazione di questa città come culla della civiltà occidentale e anche del cattolicesimo. Si tratta di aspetti che rendono Roma un *unicum* non solo dal punto di vista nazionale. L'articolo 114 della Costituzione, al comma 3, parla chiaro: affida alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento giuridico della Capitale. Dobbiamo allora constatare che, a vent'anni dall'approvazione della riforma del Titolo V, l'attuazione di questa disciplina è stata alquanto lacunosa, tormentata e sicuramente non pienamente idonea a definire uno statuto adeguato per Roma. Restano irrisolte molte questioni: la disponibilità di idonei finanziamenti, l'ammodernamento delle infrastrutture, il tema delle periferie, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche la riorganizzazione dei servizi di area vasta. E allora oggi, peraltro nel 150° anniversario della proclamazione di Roma come capitale d'Italia, esistono ragioni che rendono ancor più stringente e non rinviabile la necessità di riprendere questo percorso. Individuo due questioni: da un lato, l'approvazione del Piano nazionale che l'Europa ha messo a disposizione, le cui misure possono e debbono essere declinate in sede attuativa in modo da intercettare le esigenze e le istanze della Capitale; dall'altro, un appuntamento molto atteso, come quello del Giubileo del 2025. Di tali questioni ed esigenze il Governo è pienamente consapevole; l'intervento normativo che abbiamo in animo non può che essere multidimensionale e quindi riguardare l'architettura istituzionale, i poteri e le risorse. Questo intervento dovrà certamente allineare Roma ad altre altre capitali, tutte invariabilmente munite di statuti e poteri peculiari. In questa prospettiva, abbiamo istituito nel corso delle settimane presso il Ministero una commissione, presieduta dal professor Marini, con il compito di analizzare gli scenari di riforma dell'ordinamento di Roma Capitale, a partire dal lavoro svolto dalle Camere sulle proposte di iniziativa parlamentare. auspico e confido che ci possa essere una convergenza importante con il lavoro che il Parlamento sta facendo, in particolare la Commissione affari costituzionali della Camera, dove

quello di sostituire o scavalcare l'attività parlamentare; essa anzi aspira ad affiancarla e supportarla, con l'intento di facilitare la necessaria sintesi fra le diverse posizioni, per addivenire in tempi rapidi alla soluzione tecnicamente più adeguata per andare incontro alle esigenze di Roma e alla questione che viene posta. La commissione sta lavorando alacremente, facendo sintesi di iniziative molteplici di riforma costituzionale, ma anche di riforma ordinaria presenti in Parlamento, e della preziosa istruttoria già svolta attraverso molteplici audizioni dalla I Commissione della Camera. Vi è una sostanziale condivisione dei punti centrali di un intervento riformatore, che non può non riguardare, anche in attuazione dell'articolo 114 della Costituzione, i poteri e gli ambiti materiali delle funzioni di Roma Capitale, i meccanismi e le sedi di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, il ruolo dei municipi, le forme e le modalità di attribuzione delle risorse. La commissione si è data un termine; termine; entro fine mese mi auguro di essere in grado di illustrare le conclusioni e quindi la proposta di riforma della *governance* della Capitale. Il clima di concordia e la determinazione della I Commissione della Camera legittimano un ragionevole ottimismo sul prosieguo. Il Governo, nel rispetto delle prerogative delle Camere, monitorerà gli sviluppi dei lavori, auspicando una definizione la più celere possibile e riservandosi ovviamente di valutare ogni ulteriore iniziativa che possa accelerare l'*iter* della riforma e ampliarne gli orizzonti.

perdonatemi, ma Roma merita veramente un'altra gestione amministrativa. Tornando all'interrogazione, sono molto soddisfatto, perché il nostro sogno è quello di portare a Roma l'Agenzia della cultura europea. Roma deve diventare, anche se lo è moralmente,

Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, le immagini divulgate relative all'incidente della funivia Stresa-Mottarone lasciano senza fiato e fanno davvero male,

Il diritto di cronaca non può entrare nel dolore delle persone. Quello a cui stiamo assistendo è un tipo di giornalismo macabro e spregiudicato, che oltrepassa ogni limite e ogni logica. Il vero giornalismo è tutt'altro. I veri giornalisti sono coloro che informano i cittadini, senza toni forti, speculazioni e strumentalizzazioni. Il sensazionalismo e il *gossip* della notizia a tutti i costi non sono giornalismo, ma soltanto un modo alternativo di fare spettacolo, un vero e proprio circo mediatico, cinico e crudele, che manca totalmente di rispetto, di buonsenso e di sensibilità.

solo così si può garantire ai cittadini un'informazione degna di questo nome. Intanto, chi ha trasmesso le immagini di quei drammatici momenti si vergogni e chieda scusa.

l'Associazione nazionale vittime delle marocchinate è un sodalizio senza scopo di lucro composto da liberi giornalisti, ricercatori, storici e scrittori che da anni studiano specifiche vicende accadute nel periodo 1943-1944 in Sicilia, Campania, Lazio e Toscana, dove uomini e donne subirono violenze inenarrabili da parte delle truppe coloniali francesi, i cosiddetti *goumier*. La tragedia nazionale è passata alla storia con il termine marocchinate, che qualcuno ancora non conosce o non vuole riconoscere. L'intento dell'associazione è proprio promuovere il ricordo della storia, perché vengano condannati tutti gli errori e orrori e perché non si ripetano mai più. È purtroppo evidente che il libero lavoro degli storici venga considerato come un fastidioso e inopportuno impegno, perché ha connotazione politica. Il termine marocchinate non è inteso come razzista: era già in uso nel 1946, per cui già la sola parola non deve turbare la sensibilità ipocrita e ignorante. Così, venerdì 11 giugno 2021, a Milano, nell'aula consiliare comunale, l'associazione aveva organizzato uno dei tanti convegni dal titolo «Marocchinate: la storia nascosta», condotto alla presenza non di politici, ma di Emiliano Ciotti, presidente dell'Associazione vittime delle marocchinate, di Alessandra Colla, scrittrice e storica, e del moderatore Lorenzo Cafarchio, delle Edizioni Altaforte. Il sindaco Sala, con un *post* sui *social*, ha definito l'incontro pubblico come inutilmente provocatorio. «La storia è una cosa seria: usarla per provocazioni dal sapore di razzismo»... «è una cosa che Milano e i milanesi non possono accettare». Ovviamente il *post* è stato amplificato da vari esponenti politici, come il capogruppo del PD in Comune, che ha dichiarato: «La Lega, a corto di argomenti per la campagna elettorale, non trova di meglio che promuovere e sostenere un evento dal chiaro significato razzista». Un altro deputato del PD ha tacciato lo stesso evento come sceneggiata propagandistica di stampo razzista. Alla fine, l'autorizzazione già concessa è stata ritirata e il convegno è stato Vorrei far presente che le marocchinate non sono una bandiera politica. Vorrei far presente che non si né di destra, né di sinistra davanti a una commemorazione di vittime, soprattutto se incolpevoli. Vorrei far presente altresì che è dovere di ogni cittadino e soprattutto del politico onorare vittime innocenti: 60.000 uomini, donne, anziani, preti e bambini sono stati vittime di violenze sessuali spregianti e mortali perpetrate dai *goumier*, uccisi anche solo per aver cercato di difendere la vita di sorelle, spose e madri. Questa è la storia, che dev'essere ricordata senza la becera ipocrisia della politica scorretta;

A Sala dico soprattutto di chiedere scusa a Milano, ai milanesi e, per la sua ignoranza, a tutte le vittime innocenti di un tragico passato storico. Signor Presidente, il 14 agosto 2018 crollava a Genova il ponte Morandi, causando 43 vittime, centinaia di sfollati e gravissimi disagi per la città di Genova, la Liguria intera e l'intero Nord-Ovest del nostro Paese, oltre a un danno per l'immagine dell'Italia all'estero. In questi giorni, si è pericolosamente vicini alla conclusione di una transazione, con l'obiettivo di mettere fuori i famosi Benetton dalla società Autostrade per l'Italia, mediante l'acquisto, da parte

la cosa potrebbe essere risolta molto meglio e con molto meno. Infatti, anziché cambiare gli azionisti di una società che comunque non è lo Stato (per quanto lo Stato, attraverso Cassa depositi e prestiti vi partecipi),

calcoli), dando ancora una montagna di soldi ai Benetton, sarebbe illogico comunque, perché i regali lo Stato li deve fare a chi ne ha bisogno e non ai miliardari. Inoltre, dopo quello che è successo, è assolutamente inaccettabile.